questo decreto-legge nasce per il vivo allarme suscitato dalla diffusione della notizia della circolazione di *dossier*, intercettazioni illegali e così via. Con encomiabile sollecitudine il Governo, acquisito il consenso - a quanto si è appreso dalla stampa - dei principali *leader* dell'opposizione, ha predisposto un provvedimento finalizzato a tre obiettivi: il primo è quello di provvedere alla distruzione di questo materiale illegale onde impedire diffusione di veleni e di altri e di altri elementi di inquinamento della vita pubblica; il secondo riguarda la previsione di una nuova fattispecie di reato, legata alla detenzione del predetto materiale; il terzo punto è l'introduzione di una efficace o presunta efficace forma di sanzione nel caso di divulgazione divulgazione a mezzo di stampa o del sistema radiotelevisivo di questo materiale. Nell'attento esame che si è svolto in Commissione si è cercato di inquadrare questa normativa per più aspetti originale ed innovativa nel nostro sistema tenendo anche conto del conforme parere espresso - che ci ha incoraggiato in questa direzione - dalla Commissione affari costituzionali, di rendere coerente questa normativa al nostro sistema costituzionale e giuridico, senza impedire di produrre la sostanza degli effetti positivi che il Governo si prefiggeva. È evidente, infatti, che un sistema giuridico vive del delicato bilanciamento di interessi e valori costituzionali che, a volte, possono apparire confliggenti: la libertà di stampa da una parte e la tutela della riservatezza dall'altra; l'esigenza di evitare la diffusione di notizie false e infondate da una parte e dall'altra, tuttavia, la necessità di rispettare regole e princìpi, che a volte hanno fondamento costituzionale, in materia di tutela della collettività contro possibili reati, di garanzia della formazione delle prove e delle decisioni in sede di contraddittorio. La Commissione ha pertanto esaminato quelli che ci sono sembrati i punti di criticità del provvedimento a tale riguardo e propone una nuova, integrale riformulazione del testo del Governo che - ripeto - a nostro avviso soddisfa le esigenze fondamentali per le quali il provvedimento era stato predisposto e, tuttavia, le rende, a nostro giudizio, coerenti con i principi anche costituzionali del sistema: in particolare, il principio del giusto processo e del diritto alla difesa, che richiede che le decisioni giudiziarie di notevole rilievo si formino in contraddittorio e che sia garantito il diritto alla difesa sia sia dell'imputato sia delle parti offese; il principio della obbligatorietà dell'azione penale, che richiede che davanti a notizie rilevanti di reato, almeno a fini investigativi, la notizia non possa essere distrutta e obliterata e anche, per quanto riguarda il sistema del rapporto con la stampa, un equilibrio tra la necessità di sanzionare comportamenti illeciti e quella di tutelare la libertà di stampa. Ecco il motivo per il quale la Commissione ha approvato a larghissima maggioranza, conservando anche in questo esame, in questa valutazione, negli emendamenti quello spirito di collaborazione tra maggioranza e opposizione, che già era alla base della stesura originaria del decreto. Ricordo sinteticamente le innovazioni introdotte: per quanto riguarda gli articoli 1 e 2, la distruzione non è più immediata da parte dell'autorità giudiziaria, ma richiede un previo procedimento, che ha per altro tempi rigorosamente sanciti. È abolito il divieto di utilizzare il materiale a fini investigativi, mentre rimane il divieto di altre forme di utilizzazione processuale. Per quanto riguarda l'articolo 3, che introduce una nuova fattispecie di reato, abbiamo ritenuto di chiarire innanzi tutto che il reato di detenzione sussiste dopo che sia stata dichiarata l'illegalità del materiale medesimo e ciò avviene attraverso il provvedimento di distruzione, preso dall'autorità giudiziaria, dopo il contraddittorio previsto dall'articolo 1. Si è ritenuto altresì di meglio precisare l'elemento soggettivo dell'illecito penale, sostituendo l'avverbio «illecitamente», che era stato previsto dal Governo e che aveva suscitato dubbi e perplessità di natura giuridica, con l'altro «consapevolmente», analogamente a quanto disposto da fattispecie come, per esempio, la detenzione di materiale pornografico

c'è una riformulazione dell'articolo 4, che è una norma che prevede una figura di pena privata che l'ordinamento già in qualche caso prevede (addirittura nella legge sulla sulla stampa, che risale al 1948, poco usata, ma che può essere uno strumento interessante di intervento); si è cercato di regolare meglio la procedura, si è ridotta l'entità minima della riparazione, portandola da 20.000 a 10.000 euro. Sostanzialmente, signor Presidente, onorevoli colleghi, a me pare che la Commissione abbia svolto un lavoro costruttivo, di miglioramento del testo del provvedimento, quindi ne raccomando l'approvazione da parte del Parlamento. Chiedo fin d'ora ai colleghi, naturalmente abbiano condiviso o condividano questo *iter* e non a quelli - ci sono ancora - che hanno singoli o più ampi punti di dissenso, se lo ritengono, di ritirare gli emendamenti da loro presentati, in modo da consentire un più sollecito *iter* del provvedimento. Colleghi, molto sobriamente voglio esprimere un ringraziamento al presidente Salvi e a tutta la Commissione per un lavoro che non ha sostituito l'Assemblea, ma ha trovato rilevanti punti di incontro. Poiché non sono frutti

nei mesi passati grande interesse nell'opinione pubblica del Paese. Innanzi tutto, avverto che esprimerò un punto di vista favorevole alla normativa contenuta nel decreto-legge al nostro esame, anche se non posso fare a meno di esporre alcuni rilievi, che riguardano non tanto il contenuto, quanto soprattutto le modalità con le quali il Governo ha ritenuto di affrontare l'argomento. È vero che negli ultimi mesi in Italia si è verificata una serie di situazioni

sofferenza, di persecuzione, di indegna speculazione su intercettazioni che hanno riguardato varie persone e situazioni.

e sconcerto ed hanno provocato gravissimi danni a persone spesso assolutamente incolpevoli ed estranee. Era, quindi, naturale che nel Paese si creasse una situazione - come ho affermato poc'anzi - di sconcerto e che il Governo

Nell'ambito di tale situazione, si ebbe un momento di particolare significato quando anche intercettazioni illegalmente acquisite - come quelle di Telecom - cominciarono a dar luogo a vive preoccupazioni

però, non implicava che il Governo potesse affrontare solo questo argomento, rimandando il resto delle considerazioni, su cui il Paese chiamava

al decreto-legge. Ora, mettendo da parte queste osservazioni, che - ripeto - rappresentano le mie perplessità, dico perché sono favorevole al decreto-legge in questione. Non c'è dubbio che la materia va rivista tutta, interamente, e che danni

inopportunamente utilizzate. Se, però, su questo non c'è stata sufficiente attenzione e sensibilità, ciò non esclude che il segnale

rimedia ad una lacuna legislativa - che anche comportamenti che si affiancano all'illecita acquisizione di conversazioni telefoniche (come la detenzione o l'utilizzazione delle stesse) sono comportamenti

dei cittadini e questa utilizzazione del congegno delle intercettazioni limitata e codificata ancora meglio rappresentano certamente un fatto positivo. Questa - ripeto - è la ragione per la quale condivido il decreto‑legge.

attraverso una serie di emendamenti che verranno illustrati successivamente. Il nucleo fondamentale è quello di provvedere, nel più breve tempo possibile, alla distruzione di queste intercettazioni. Una distruzione che è determinata da un desiderio: l'esigenza che venga meno lo strumento che può dar luogo a quelle gravissime conseguenze per la *privacy* e la tranquillità dei cittadini. Concludo ribadendo che, per tutte queste ragioni, sono favorevole alla conversione del decreto-legge, con gli aggiustamenti prodotti dalla Commissione; voterò quindi a favore della legge di conversione. Mantengo le mie riserve per un'importante occasione che il Governo si è lasciato sfuggire. Mi auguro che al più presto la Camera, che in questo momento si sta occupando di rivedere la disciplina delle intercettazioni, faccia in modo, affrontando la tematica complessiva delle intercettazioni, che non soltanto i cittadini che sono stati toccati in qualche modo dalla vicenda Telecom, ma anche le altre centinaia, migliaia o milioni di cittadini italiani possano trovare al più presto una rapida ed efficace tutela.

operato sotto la spinta di eventi che hanno colpito in maniera pesante l'opinione pubblica di questo Paese e che hanno destato giuste preoccupazioni, disvelando attività non soltanto lesive per la garanzia della sfera della privatezza individuale, ma anche tali da porre a rischio la tenuta complessiva del sistema. Ci siamo trovati certamente ad operare in condizioni non facili che si sono poi - come è ovvio e come era probabilmente inevitabile riflesse anche sullo svolgimento dei lavori parlamentari, soprattutto considerando la necessità di salvaguardare un equilibrio sicuramente complesso, sicuramente difficile, in una materia di assoluta delicatezza

di privatezza di sicuro rilievo costituzionale: ambito e che, negli ultimi anni, ha giustamente visto accrescere la sensibilità del legislatore e dell'opinione pubblica quanto alla sua difesa. Sono in campo ovviamente gli interessi di giustizia. Una categoria che va dal rispetto delle garanzie, di cui agli articoli 24 e 111 della Costituzione, della stessa persona che venga eventualmente accusata di aver posto in essere l'illecita acquisizione di dati; agli interessi di giustizia intesi sotto il profilo del possibile ostacolo posto ad attività investigative dirette alla tutela della sicurezza pubblica e che non si concretino nell'acquisizione della intercettazione in sé, ma trovino fondamento sulle

Sarebbe, con ogni evidenza, troppo facile - se si desse una soluzione squilibrata - che il malfattore organizzasse a proprio danno l'intercettazione illecita per trarre poi da questa un comodo

Sono convinto della incostituzionalità dell'attuale formulazione dell'articolo 4. Mi dicono adesso che c'è stata una modifica apportata in Commissione. Se va nel senso che dirò, me ne compiaccio davvero vivamente. Sono convinto dell'incostituzionalità dell'attuale formulazione perché con la formula utilizzata - la divulgazione degli atti o documenti - noi colpiamo la stampa non soltanto per la pubblicazione della trascrizione. Per fare un esempio, non solo perché si pubblica «Tizio dice, Caio risponde», ma anche per la diffusione di notizie concernenti l'intercettazione.

a mio avviso, la giusta luce su situazioni portate all'attenzione della pubblica opinione. Mi rendo conto che probabilmente non abbiamo la migliore stampa del mondo; questo lo dico anch'io.

punisce la detenzione del documento o dell'atto, non sono d'accordo e ritengo incostituzionale l'articolo 4, che usa una formula troppo generica.

all'esame dell'Aula, dopo una serie di turbolente questioni che l'hanno sempre accompagnata, è utile per cercare

allora tentarne una lettura, signor Presidente, che parta da quello che è il vero problema, del quale nessuno parla. Il problema non è tanto come regolamentare le intercettazioni legali: il problema reale è la vicenda Telecom. In un Paese democratico come il nostro, dove è prevista una magistratura il cui intervento è sempre puntuale rispetto alle vicende che determinano

Questa è la prima domanda che dovremmo porci, altrimenti stiamo discutendo di qualcosa che non riusciremo mai a comprendere fino in fondo.

non è stata oggetto di questo decreto-legge, ma di un disegno di legge che è stato presentato e giace alla Camera. Il decreto-legge che è stato sottoposto all'esame

era un'iniziativa truffaldina dedicata a controllare i Palazzi; o a servirli, perché probabilmente vi era anche qualche Palazzo che si serviva di questa rete parallela, di questo fiume carsico di notizie che attraversava la nostra beneamata Repubblica. Questo è un altro dato del quale non parliamo, diciamo che stiamo varando delle norme che servono ai cittadini: non è vero! Le norme che servono ai cittadini sono quelle che in questo momento sono state presentate nell'altro ramo del Parlamento, alla Camera. Esse riguardano tutti quei soggetti che hanno la sfortuna di incappare in intercettazioni legali, non illegali come queste, l'utilizzazione delle quali viene distorta e che quindi finiscono sui *mass* *media*, sulla stampa e diventano note. In questa sede trattiamo invece questioni completamente diverse. Poco fa il senatore Andreotti

tutte quelle che vengono fatte fuori da un sistema che in Italia prevede assolutamente sempre il controllo della magistratura. questo tipo di deviazione relativa alle intercettazioni che passano dalla magistratura, si occupa la Camera; al Senato ci occupiamo di un'altra fattispecie. Se partiamo da questo dato, comprendiamo il perché di certi accadimenti che si sono succeduti in questi giorni e la necessità di chiudere una vicenda eccezionale. Il «dossieraggio» operato dalla Telecom è una vicenda inquietante, che funesta la nostra democrazia? Certamente sì! Una questione eccezionale, non ordinaria, non routinaria? Certamente sì! Proprio per questo,

mentre altre non passano, nella quale affermo: «Il decreto-legge del Governo è inapplicabile». Era inapplicabile, Presidente, ed è, secondo me, in parte ancora inapplicabile perché perché non si inserisce in un contesto nel quale si verifichi qual è realmente la posta in gioco, cioè la riservatezza, calandola in un mondo fatto di valori e di esigenze e rendendola compatibile con tutto il resto. La riservatezza è un valore? Sicuramente sì. L'obbligatorietà dell'azione penale è un altro valore che si deve coniugare e comparare con la riservatezza? Certamente sì. L'articolo 111 sul giusto processo, quella conquista che nella 13a legislatura tutti abbiamo condiviso, è un altro valore?

avesse deciso di immettere nel nostro sistema questa anomalia. Tale anomalia, anziché contemperare le varie esigenze, i princìpi, le conquiste ed i valori della nostra civiltà giuridica, operava una scelta. In questo caso,

se vogliamo tentare di correggere quel decreto-legge, che nasceva però con l'aspirazione di compiere una scelta che tenesse parzialmente conto dell'eccezionalità della vicenda, ma non era obiettivamente condivisibile in un panorama complessivo.

per la gente comune. Questa era una vicenda di palazzo, un palazzo ampio composto di maggioranza e opposizione, di potentati e signorie.

Signor Presidente, con la necessaria tempestività, e con l'accordo dell'opposizione, il Governo ha emanato il 22 settembre scorso un provvedimento d'urgenza finalizzato ad individuare misure idonee a rafforzare il contrasto all'illegale raccolta e detenzione di contenuti, dati, documenti e informazioni relative al traffico telefonico dei cittadini, prevedendo, al contempo un intervento più incisivo per evitare l'indebita diffusione e pubblicazione di dati o elementi illegalmente acquisiti.

77 della Costituzione pone quali requisiti insormontabili per l'attribuzione al Governo del potere di emanare atti aventi immediatamente forza di legge. Requisiti che devono essere ancor più stringenti se, come in questo caso, si incide sulla libertà personale, sulla qualificazione di alcuni comportamenti come reato e sulle modalità di esercizio di diritti costituzionalmente garantiti. Da molto tempo l'incessante pubblicazione di stralci ed estratti di conversazioni telefoniche, oggetto di intercettazioni, regolarmente disposte dall'autorità giudiziaria e la divulgazione anche integrale di atti processuali coperti da segreto o comunque da vincolo di riservatezza, ha posto al centro del dibattito politico la necessità di una riflessione su come garantire il contemperamento di alcune libertà costituzionali (a cominciare dal diritto di cronaca e dal diritto ad essere informati) con l'esercizio di altri diritti costituzionalmente rilevanti, quali ad esempio il diritto alla difesa, la tutela della dignità della persona e la salvaguardia dei dati sensibili personali. Tutti hanno convenuto sull'esigenza di assicurare, con efficacia e su un piano generale, un'adeguata tutela dei diritti delle persone coinvolte dalla pubblicazione di innumerevoli brani di conversazioni intercorse anche con terzi, estranei ai fatti oggetto di indagine penale, o che non risultano allo stato indagati, o brani che riguardano in ogni caso diverse relazioni personali o familiari o, ancora, persone semplicemente lese dai fatti. Abbiamo assistito anche alla pubblicazione di conversazioni riguardanti comportamenti strettamente personali di persone pur coinvolte nelle indagini, ma non direttamente connessi a fatti penalmente rilevanti. Tutto questo è da tempo al centro del dibattito politico: anzitutto dalla magistratura, ma anche dagli operatori dell'informazione e del diritto, sono venute indicazioni preziose per affrontare questi temi, evitando l'onda dell'emozione, che spesso induce a modifiche affrettate e poco meditate come quelle proposte nel dicembre 2005 dal Governo Berlusconi, le quali avrebbero avuto, se approvate, il solo effetto certo di danneggiare irreparabilmente l'attività di indagine dei magistrati e di rendere difficile, se non impossibile, per l'opinione pubblica la conoscenza di situazioni e fatti di indubbio rilievo. Quello che invece è emerso più recentemente, in tutta la sua vastità, è un fenomeno ben diverso e ben più inquietante. È stata svelata, grazie ad una lunga e difficile indagine, una attività del tutto illegale, posta in essere da alcuni soggetti che, utilizzando strutture e mezzi tecnologicamente avanzati, in virtù degli uffici e delle funzioni da essi ricoperte in uno snodo particolarmente delicato del sistema delle comunicazioni, avrebbero costituito nel corso di almeno un decennio una raccolta imponente di dati, documenti, informazioni e (forse) anche contenuti del traffico telefonico di migliaia di cittadini. Il tutto, va ripetuto, è accaduto ad di fuori di ogni previsione di legge e al di fuori di qualunque ambito di indagine giudiziaria. Le caratteristiche della struttura aziendale nella quale costoro avrebbero operato e la vastità del sistema illegale da essi messo in piedi possono a ben diritto farci dire che mai ci si è trovati di fronte ad un fenomeno così ampio e grave di violazione dei diritti personali. All'interno o comunque nell'orbita diretta o indiretta della più grande azienda italiana di telecomunicazioni, che peraltro si è dichiarata estranea ai comportamenti degli indagati e si è costituita parte lesa, avrebbe operato, per usare i termini dell'ordinanza di custodia cautelare del Gip di Milano, «una vera e propria ragnatela parallela» in grado di usare «tutti i mezzi concretamente esistenti sul mercato» per raccogliere «qualsiasi tipo di informazione», violando «i princìpi costituzionali fondanti di questo Paese». Gli «spiati» sono soprattutto imprenditori e finanzieri, ma i *file* illegali sarebbero più di centomila e coinvolgerebbero dipendenti, possibili concorrenti e avversari persone influenti da «tenere eventualmente in pugno», con tanto di «accessi abusivi al sistema dell'anagrafe tributaria» e agli archivi bancari. La compravendita clandestina di tabulati telefonici si sarebbe affiancata persino all'acquisto di notizie riservate sulle banche dati dell'Interno, dell'Economia, della Giustizia, comprendendo «informazioni e atti svolti da agenti e pubblici ufficiali». Questa enorme massa di informazioni illegali e di dati riservati sarebbe stata commissionata e pagata da un manipolo di persone che non risultavano soggette ad alcun vero controllo. Questo è il quadro di un sistema illegale che ha attentato, secondo i magistrati, ai diritti di migliaia di persone, a cominciare da operai e dipendenti, ed addirittura da aspiranti dipendenti (cioè da coloro che avevano presentato la loro domanda di assunzione); in questo senso non condivido il riferimento al fatto che queste indagini non si riferiscano a gente comune: gli operai, i dipendenti sono gente comune. Ad aggravare il quadro, contribuisce certamente il sospetto investigativo che la raccolta illegale dei dati avvenisse a scopo di lucro, per farne illecito commercio, per trarre profitto dalla divulgazione o dalla minacciata divulgazione di questi atti, oppure con la finalità di tenere sotto controllo i movimenti ed i contatti delle persone vittime dell'attività illegale. Allo stato degli atti, noi non sappiamo chi e perché abbia effettivamente ordinato la raccolta dei dati, quale uso ne sia stato eventualmente fatto e se, ad esempio, sia stata avviata un'attività di «dossieraggio» che per ampiezza e gravità supererebbe perfino le ormai antiche schedature del SIFAR o per altri versi quelle famose della FIAT degli anni Settanta (schedature che, voglio ricordare, hanno riguardato tutti i dipendenti del gruppo FIAT e tutti gli aspiranti dipendenti del gruppo FIAT). Ciò è oggetto di indagine e su questo si pronunceranno i giudici. Quel che oggi è certo è che una mole imponente di dati è stata illegalmente raccolta dal 1997 ad oggi. E questo di per sé basta a far temere che alcune libertà fondamentali siano state messe a rischio. Sulla base degli atti che emergono nell'ambito delle indagini preliminari in corso presso gli ufficio giudiziari, le ipotesi di reato in fase di accertamento denotano circostanze per le quali è indubbio un interesse pubblico e che fossero urgentemente prescritte regole capaci di stroncare l'illecito trattamento dei dati telefonici, prevenendo il rischio che da questa pratica si sprigionasse un'incontrollabile nuvola di informazioni velenose. Una rapida scorsa alle 344 pagine dell'ordinanza di rinvio a giudizio lascia sgomenti: il numero delle persone coinvolte è altissimo. Il decreto intende affrontare questo rischio e parte dal presupposto che certo nessuna norma e nessun controllo possono annullare del tutto il rischio più grave, quello che siano proprio gli addetti alla sicurezza dei dati a violare la sicurezza. Per questo si è voluto, oltre alle previsione di forti sanzioni, assimilare al trattamento già previsto per i documenti anonimi gli esiti delle intercettazioni illecitamente effettuate e dei dati relativi al traffico telefonico Va in questo senso la decisione di procedere alla distruzione da parte dell'autorità giudiziaria di tutti gli atti e i dati acquisiti ovvero anche solo illecitamente detenuti. Questi sono i due elementi centrali del decreto e con il lavoro del Parlamento sul testo e le modifiche e i miglioramenti apportati è ragionevole pensare, ad esempio, che sia il giudice a disporre la distruzione, assicurando il contraddittorio fra le parti oppure consentire che il corpo del reato possa comunque costituire spunto di indagine, in modo da non comprimere né il diritto alla difesa né l'obbligo costituzionale all'esercizio dell'azione penale. Noi pensiamo, che la detenzione vada punita qualora si intenda pubblicare o fare uso illecito di questi dati da parte del detentore. Riteniamo inoltre importante non comprimere in alcun modo il libero esercizio dell'attività giornalistica, anche perché va ricordato

di un provvedimento dei paradossi e dei misteri. Il paradosso è che il Governo in tutta fretta vara un decreto-legge, quindi una norma che contiene

non vi è alcuna indagine in corso su questo tema. In questo paradosso cade anche il collega che mi ha preceduto, il quale è convinto

che sono state svolte da personaggi che possedevano anche agenzie di investigazione in maniera, a quanto pare, illegittima. Ma si parla di indagini e di acquisizione di dati, non di intercettazioni. Questa è la prima questione che va evidenziata. Se vi sono, poi, indagini coperte da segreto, questo ovviamente non possiamo saperlo, ma al momento, ufficialmente, non esiste alcuna indagine che abbia individuato come fattispecie di reato l'acquisizione illegittima relativa alle intercettazioni telefoniche o telematiche. Il paradosso è che il Governo interviene addirittura con un decreto-legge su questo tema. Interviene sul nulla.

ripeto: 1 miliardo e 200 milioni di vecchie lire per ogni seduta che apriamo al Senato. Forse varrebbe anche la pena di impiegare in maniera ottimale il denaro dei contribuenti. è poi il mistero, perché all'atto del varo di questo decreto il Presidente del Consiglio ha dichiarato che il decreto-legge varato dal Governo sulle intercettazioni - quindi non sulle indagini - nasce per evitare

Che cosa sa per essere indotto a varare in tutta fretta un decreto che - si badi bene - se l'avessimo proposto noi, nel precedente Governo, con la precedente Presidenza della Repubblica, non avrebbe mai ottenuto la firma da parte del presidente Ciampi, perché mai su una materia del genere avrebbe ravvisato la straordinaria urgenza? Prova ne che, quando abbiamo voluto fare un decreto su questa materia, siamo stati «stoppati» e abbiamo dovuto fare un disegno di legge. Il secondo paradosso è ciò che è accaduto ieri: il Governo

Improvvisamente ieri - non so se cronologicamente ciò è importante, ma dopo che in mattinata l'ANM è stata accolta in dialogo, in discussione con il Presidente del Consiglio - il Ministro della giustizia, senza nemmeno avvisare la maggioranza, presenta un emendamento che di fatto è un nuovo decreto e che ribalta in maniera copernicana l'impostazione del primo testo. Nel primo testo le intercettazioni devono essere immediatamente distrutte, nel secondo testo devono essere distrutte dopo che una sentenza di un procedimento penale è passata in giudicato, cioè dopo dieci anni, cioè di fatto mai. Questo è il secondo grave paradosso a cui segue il terzo, perché dopo altre due ore il Governo ci ripensa un'altra volta, ritira l'emendamento e si torna al decreto, al testo precedente. Allora qui, evidentemente, c'è un altro mistero: perché è stato fatto ciò, quali sono i motivi, quali sono le ragioni? Silenzio. Soltanto silenzio da parte del Governo, perché non si può dire che si sia cercata una mediazione: non è una mediazione ribaltare in maniera copernicana il testo di un precedente decreto-legge (che, ripeto, è urgente, inderogabile e quindi necessario: stiamo parlando non di un disegno di legge, ma di un decreto-legge), poi cambiare totalmente e dopodiché cambiare ancora. Vogliamo sapere la ragione, quali sono stati gli eventi esterni all'Aula che hanno portato a ciò. Su questo non ci è stata data alcuna spiegazione, ma devo dire anche che nessuna spiegazione è stata richiesta se non, forse, in questo momento. Ebbene, credo che il Governo abbia il dovere di dire esattamente che cosa è accaduto.

stiamo lavorando su dei testi che, di volta in volta, sono esattamente il contrario di quello che ci è stato presentato qualche ora prima. Infine, un ultimo paradosso: questo decreto non va a toccare minimamente il problema vero e reale del cosiddetto scandalo delle intercettazioni che avviene nel nostro Paese, cioè la propalazione di queste ultime sui giornali e sui *media*. Ricordiamoci che questi cosiddetti scandali nascono tutti da intercettazioni che sono state legittimamente acquisite, attraverso ordinanze della magistratura. Dunque, è illegittimo l'uso, cioè la propalazione di queste intercettazioni, alcune volte violando il segreto istruttorio, quindi commettendo un reato, altre volte non ottemperando alle previsioni di legge, alle previsioni normative del codice di procedura penale, depositando atti che in quel momento evidentemente diventano pubblici, ma che contengono stralci di intercettazioni che magari nulla hanno a che vedere con l'inchiesta in corso e che servono soltanto, alcune volte a colpire delle persone, altre volte a soddisfare la sete di *gossip*

che è meramente virtuale, che agisce su un'attività meramente virtuale, di cui noi non abbiamo fino adesso alcuna prova. Questo è l'ambiente in cui, al momento, ci apprestiamo a lavorare. Per cogliere l'occasione (perché questa è veramente un'occasione perduta, dato che si rinuncia a intervenire su quello che è invece il tema reale, l'uso illegittimo di intercettazioni acquisite legittimamente), noi abbiamo presentato una serie di emendamenti che mi riservo di illustrare.

durante i lavori di Commissione, si sono confrontate ipotesi diverse: vi è stata certamente una dialettica serrata, ma apprezzabile, se è vero, com'è vero, che si è giunti ad ipotizzare una soluzione per larghi versi condivisa. E non poteva essere diversamente, attesa la materia che si stava trattando e le ragioni che avevano indotto la trattazione così sollecita, così celere: l'adozione dello strumento del decreto; una materia resa incandescente, se mi si passa l'espressione, proprio dalla vicenda Telecom che aleggia in quest'Aula, della quale si parla poco, di cui poco si è parlato anche quando il Presidente del Consiglio è venuto a riferire di temi correlati. Abbiamo avuto la sensazione di quanto precaria sia la *privacy*, la riservatezza alla quale ognuno ha diritto, come, attraverso questi strumenti della modernità, usati in maniera perversa, si possano realizzare attività intrusive per entrare ad esempio nelle case di soggetti che non debbono

in sintonia con il sistema: viviamo in uno Stato di diritto, lo ripetiamo sempre per ricordarlo a noi stessi gli strumenti che dobbiamo adottare debbono essere in assoluta sintonia con il sistema viviamo. Ebbene, al di là delle osservazioni ulteriori che certamente nell'ambito della trattazione in Aula saranno fatte, credo che il prodotto finale che la Commissione ha realizzato sia tutto sommato apprezzabile. Devo dare atto - lo faccio perché me lo impone l'onestà intellettuale - al Governo di aver ritirato un emendamento presentato in un contesto le cui connotazioni precise ancora ci sfuggono; un emendamento che avrebbe alterato lo spirito del decreto, la filosofia, le ragioni

coronati da un successo sostanziale, diciamolo pure. Il Presidente del Senato ha capito l'importanza dell'impegno; ci ha consentito una trattazione nel corso della mattinata di oggi senza pressioni di alcun genere;

sono particolarmente interessato e che pongo in questa fase di discussione generale, anche se il senatore Storace lo tratterà partitamente: è quello relativo allo spionaggio politico e alla cesura di provvidenze ai politici che pongano in essere attività connotate da questo tipo di illiceità. Io non so quale quale strumento si possa adottare per superare l'eventuale sbarramento che, attesa la trattazione del tema, la maggioranza qualificata impone; tuttavia, ove mai il voto fosse corale, sarebbe votato con maggioranza qualificata, dunque potrebbe introdursi nel decreto anche l'emendamento 4.0.1, al quale tutti noi teniamo, a riprova che vi è una parte politica in questo Paese che non chiede guarentigie particolari per chi siede nei banchi del Parlamento, per chi sta nel Palazzo, come diceva poc'anzi il

Signor Presidente, ritengo che le intercettazioni siano uno strumento importante - parlo di questo segmento delle attività intrusive che si svolgono nell'ambito dell'esigenza processuale - e che siano indispensabili per la realizzazione delle finalità che il processo persegue, per accertare responsabilità, per accertare verità. L'uso che da qualche tempo se ne fa è un uso perverso; le intercettazioni sovente vengono fatte per essere sbandierate sui giornali, prescindendo dagli esiti che si realizzeranno nell'ambito del processo. Che siano serventi al processo è un fatto quasi marginale e ciò che io lamento, signor Presidente, lo dico con amarezza, è che molto spesso inutili intercettazioni vengono regolarmente disposte, assolutamente ininfluenti rispetto alle esigenze processuali, soltanto per poterle depositare, per poterle ufficializzare e perché siano divulgate non per l'importanza che esse hanno nell'ambito dell'esigenza processuale, ma perché alcuni contenuti suggestivi possono suscitare turbamenti, climi particolari,

che ha suscitato grande clamore per la qualità dei protagonisti: quella relativa alle intercettazioni UNIPOL, atti che, al di là dei fatti e della rilevanza politica, dei quali non è il caso di parlare in questa sede perché in questa sede certamente non ci interessano, erano stati destinati allo stralcio, alla cancellazione, alla soppressione, e che sono stati poi utilizzati in maniera clandestina e spregiudicata. Ebbene, credo che chi si rende responsabile di condotte di questo genere debba pagare adeguatamente e il decreto anche questo prevede. Interventi, quindi, per cancellare l'oggetto delle nefandezze, censure rigorose per coloro che sono protagonisti, che sono responsabili di queste nefandezze. Francamente, altro strumento non vi era, se non quello del decreto, per porre argine a questo stato di cose. Che si discuta nell'altro ramo del Parlamento un disegno organico teso a rivisitare questa complessa materia è fatto certamente apprezzabile, del quale assumeremo cognizione quando si trasmetterà il testo in questo ramo del Parlamento e al quale daremo i contributi necessari secondo le esigenze le esigenze che avvertiamo e che riteniamo debbano essere coerenti con le principali esigenze della giustizia. Credo, signor Presidente, che il Senato possa compiere questo ulteriore sforzo per esaminare gli emendamenti: alcuni meritano di essere considerati con la massima attenzione, affinché in tempi celeri il provvedimento possa essere licenziato. Certamente, Alleanza Nazionale non farà mancare il proprio contributo. Presidente, quando è iniziata la trattazione del disegno di legge in esame, mai avrei immaginato di intervenire in sede di discussione generale.

le stranezze che ne hanno accompagnato l'*iter* (da ultimo quello *stop and go* che ha caratterizzato la giornata di ieri, con l'emendamento del Governo), mi impongono di intervenire, per rappresentare all'Aula talune mie perplessità. Ho ascoltato gli interventi del senatore Manzione e, da ultimo, del senatore Valentino. Trovo davvero singolare che, a fronte di anni e anni di macelleria mediatica, che ha trovato il suo presupposto proprio nell'indebita e reiterata fuga di notizie, portando all'infangamento di moltissime persone, il Governo abbia deciso di intervenire, con un decreto‑legge, con riguardo ad un episodio come quello della Telecom, ma assolutamente marginale rispetto all'incredibile ed intollerabile fenomeno che ha caratterizzato la vita, non solo politica, di questi ultimi anni. Si ritiene che vi siano ragioni di necessità e urgenza in considerazione di quanto accaduto nell'episodio di «spionaggio» Telecom. Bene: nel corso dei lavori della Commissione abbiamo appreso, però, che in quello spionaggio non vi è stata nessuna intercettazione telefonica e che il tutto si è limitato ad un'acquisizione illecita di taluni tabulati di traffici telefonici,

ha affermato di essere stato vittima dello spionaggio della Telecom. E così, ci troviamo di fronte ad un decreto‑legge emesso, per necessità e urgenza,

di nuovo al testo originale che, però, sappiamo sarà modificato, in ragione degli emendamenti a firma della Commissione, poiché è stato raggiunto un accordo. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non credo che il tecnicismo, che pure a volte dovrebbe accompagnare le norme, sia di per sé utile alla risoluzione dei problemi politici; spesso, però, questo, se male utilizzato, svela svela i reali obiettivi che attraverso una norma si intendono raggiungere. E diciamolo francamente: l'obiettivo che si intendeva raggiungere fin da subito non era e non è la tutela dell'immagine e della *privacy* dei cittadini italiani, troppo a lungo vulnerata dalla macelleria mediatica, ma era semplicemente la necessità di tutelare la *privacy* di quei ben individuati soggetti che erano stati oggetto di uno spionaggio politico, di uno spionaggio da parte della Telecom. Nell'ignoranza di quali fossero e di quali siano questi soggetti, non potendo evidentemente rientrare il calciatore Vieri in uno spionaggio della Telecom ma semmai in una forma di pedinamento, rimane - per sua stessa ammissione - come unico soggetto noto parte lesa l'attuale Presidente del Consiglio. Certo è che noi andiamo a regolamentare questo piccolo segmento dell'anomalia italiana consentendo, in ragione del fatto che alla Camera si discute di altro disegno di legge o di proposta di legge, che quotidianamente i giornali, attraverso la veicolazione di intercettazioni legalmente autorizzate destinate a restare segrete, possano continuare a infangare l'onore e la reputazione dei cittadini. Si poteva fare meglio, nel senso che fin da subito si poteva immaginare che quella distruzione dei documenti avvenisse in forma garantita e cioè che venisse assicurato un contraddittorio tra le parti, che il soggetto deputato alla distruzione fosse il giudice per le indagini preliminari. Prendo atto però che nell'emendamento della Commissione vi è, come dire, una modifica all'originario impianto e si è costruito un procedimento in camera di consiglio che comporta, nel rispetto del contraddittorio delle parti, la distruzione dei documenti. Mi permetto però di dire che secondo quell'emendamento la distruzione dei documenti è eventuale, non è un dato certo, non comprendendosi bene il significato dell'inciso: «nel caso disponga la distruzione dei documenti»; in altri termini, non comprendendosi se la distruzione dei documenti non è ordinata quando quel reato non venga considerato ipotizzabile dal giudice per le indagini preliminari, ovvero il giudice per le indagini preliminari non intenda procedere immediatamente alla distruzione per chissà quali ragioni istruttorie evidentemente correlate al reato presupposto di intercettazioni abusive. Se la mancata distruzione del documento dovesse derivare dal fatto che il giudice per le indagini preliminari non ritiene sussistenti gli elementi, i fondamenti del reato presupposto, *nulla quaestio*. Ma se la mancata distruzione dei documenti dovesse ancorarsi a malintese o presupposte esigenze istruttorie tendenti agli accertamenti del reato, se non ricordo male, di cui all'articolo 615-*bis* del codice penale, non v'è dubbio che verrebbero vanificati non solo lo scopo della norma, ma quelle ragioni di necessità e di urgenza che sono state sbandierate come essere a fondamento del decreto stesso. E ancora

vi siete posti il problema che il reato presupposto nella forma normale, cioè quella di un privato cittadino che procede ad una intercettazione abusiva, è un reato procedibile a querela di parte? a querela di parte? E avete posto alla vostra attenzione che in assenza di querela non vi è procedibilità e che in assenza di procedibilità non vi è alcuna possibilità di incardinare in via definitiva, attraverso la distruzione, il sequestro stesso, deponendo in tal senso non le povere parole di chi vi parla, ma l'articolo 14 della Costituzione? Cosa ben diversa è, senatore Di Lello - se è questo che intende con il suo dissentire - fare riferimento alla possibilità, comunque, di procedere a confisca del corpo di reato nei casi eccezionali in cui ciò è previsto, perché quei corpi di reato costituiscono di per sé illecito; penso, ad esempio, all'arma che viene distrutta. E inoltre: perché vi ostinate a immaginare che quel verbale che rappresenta le operazioni di distruzione debba essere assoggettato alla normativa di cui all'articolo 512 del codice di procedura penale, in tema di lettura debba invece - come sarebbe più logico e sensato, costituendo semplicemente l'altra faccia di un decreto di sequestro appartenere direttamente, fin dall'inizio, al fascicolo del dibattimento, costituendo così piena prova nei confronti del soggetto per ipotesi imputato del reato di intercettazioni abusive?

Vi rendete conto che questa vostra normativa consente un regime particolarmente garantito nei confronti di un tabulato di traffico telefonico, ma non consente analoga disciplina riguardo, ad esempio, alle lettere

l'articolo 25 della Costituzione e l'articolo 1 del codice penale stabiliscono il principio di legalità e tassatività, difficilmente sarà possibile un'interpretazione estensiva *in* *malam partem* nella materia che ci riguarda.

una particolare durezza sotto il profilo della disciplina processuale imponga delle tenerezze, per così dire, sotto il profilo sanzionatorio (tenerezze che, devo dire la verità, spesso appartengono alla vostra parte politica),

le sanzioni non sono tali da svolgere il loro contenuto preventivo. Rimane solo la distruzione di quei documenti,

dal buco della serratura, tutto ciò che accade nelle famiglie delle persone che hanno la sventura di essere oggetto di intercettazione telefonica. Infine, senatori Manzione e Valentino,

di un'intercettazione telefonica legalmente autorizzata che non viene reso pubblico attraverso un provvedimento di trascrizione reso dal giudice per le indagini preliminari, e che conseguentemente è destinato a restare segreto, ove mai fosse oggetto di divulgazione si assoggetterebbe a questa stessa disciplina. Questa è l'unica ragione per la quale, pur con tante perplessità,

di sanzionare in termini duri e pesanti quella macelleria mediatica alla quale tante persone perbene di questo Paese sono state assoggettate per la superficialità linguistica di agenti e ufficiali di Polizia, magistrati, giornalisti e, scusatemi tanto, nel silenzio di una classe politica che si è limitata spesso a ritenere che una determinata fuoriuscita poteva essere utile ai propri interessi di bottega.

Condivido l'affermazione del senatore Ziccone, dopo questo lavoro attento che il Parlamento sta affrontando

Questa logica della norma sulla vicenda o sul caso noi l'abbiamo sempre contrastata e la riteniamo fortemente dannosa e lesiva dell'ordinamento. In Commissione abbiamo lavorato cercando di contenere la spinta ad

o personalità rilevanti e autorevoli: riguarda, come diceva già il senatore Tibaldi, i cittadini. Intervenire su come si utilizza materiale illecito è una garanzia per i cittadini, perché i fascicoli possono essere stati costruiti anche su lavoratori dipendenti, su cittadini qualsiasi che non hanno notorietà particolare, posizioni politiche o economiche particolari o interessi specifici da tutelare. Non è compito né del Governo né del Parlamento appurare i fatti, intervenire rispetto alla consistenza di oggetti di questa o quella indagine. Noi, di fronte a tali vicende, ci siamo posti un'altra domanda e dobbiamo affrontare un altro problema: le norme che abbiamo offrono una sufficiente garanzia di ripristino e di efficacia della legalità in questa materia?

cosa, gli atti e i documenti acquisiti da attività illecite non possono in alcun modo essere utilizzati, non possono produrre effetti positivi, né per le indagini né a fini processuali; in secondo luogo, si rafforza la tutela della legalità, sapendo che sono in gioco beni costituzionali essenziali come la libertà e la riservatezza delle comunicazioni, la garanzia della *privacy*, che è un terreno aperto

e la sua efficacia, se cioè la necessità dell'intervento tempestivo, distruggendo materiale illecito, non si esponesse e non rischiasse, dal punto di vista della definizione delle nuove fattispecie di reato e delle procedure sia penali che civili contenute nel decreto, di non tutelare la legalità, in piena rispondenza ai princìpi della Costituzione in primo luogo - quelli sul giusto processo ed altri - e alla tutela dei diritti delle parti interessate, sia delle parti lese sia degli autori del reato. reato. Dare garanzia ai soggetti implicati è essenziale per chi voglia operare con decreto nello spirito e nel fine di rafforzare la tutela della legalità. Non si possono prevedere smagliature proprio su questo. su questo. Abbiamo quindi riformulato interamente il decreto, salvaguardandone le finalità e gli scopi, ma riformulando tutti e quattro gli articoli che lo costituiscono. Naturalmente, gli emendamenti elaborati insieme, con un confronto serrato, dove tanto ho appreso dalle competenze anche giuridiche di molti colleghi dell'opposizione e della maggioranza,

che uno dei punti più delicati di intervento in questa materia, non soltanto su questo decreto ma in generale sulla materia delle intercettazioni telefoniche e telematiche, sia la tutela della libertà di stampa. Nell'emendamento della Commissione abbiamo sostituito il termine «pubblicazione» con

deve essere comunque divulgata in nome della trasparenza. Questa idea di trasparenza porta a un controllo e ad una invasività nella vita, nella *privacy*, nelle libertà dei cittadini (e insisto, di tutti i cittadini, uomini e donne). Noi non possiamo accettarlo.

destinato a minare e colpire onorabilità e credibilità di persone appartenenti a molti contesti della società.

Il decreto-legge entrò in vigore e questo ramo del Parlamento iniziò doverosamente ad esaminarlo e discuterlo. Si deve alla costante presenza del sottosegretario Li Gotti

dell'esame del provvedimento, essendo a tutti noto che quel decreto-legge non interveniva in forza di un bisogno generico avvertito dal ministro Mastella, ma veniva emesso sulla base

A questo punto è iniziato l'esame degli emendamenti - mi perdonerà, signor Presidente, se salto qualche puntata per evitare di tediare lei e i colleghi

da parte dell'intera rappresentanza popolare su un argomento di particolare rilevanza. Nessuno può dire che il Ministro, muovendosi metodologicamente in questa direzione, non abbia compiuto qualcosa che sia in sé condivisibile e non, semplicemente, quello che oggi va sotto la denominazione di politicamente corretto, ma abbia sostanza e meritevolezza. Salto le puntate successive: quando la maggioranza, entrando nel concreto degli emendamenti, delle proposte di modifica, dell'esistente e delle parti da modificare, sta per raggiungere un consenso complessivo e sta per portare la sua proposta politica e legislativa alla Commissione, succede un fatto assolutamente straordinario, anzi due. Il ministro Mastella ieri, verso la metà della mattina, annunciato a tutti che il decreto-legge non si modificherà neanche di un vocabolo, che egli non sottostà al consueto ricatto del suo solito collega di Governo, del solito Ministro che gli è concorrente,

oggi l'Assemblea del Senato voterà. Verrebbe da esclamare, e se lei crede forse lo posso fare a conclusione del mio intervento, che tutto è bene quel che finisce bene.

Cercando di non urtare gli scogli che intralciano la navigazione a destra e a sinistra, oppure tentando di accontentare l'uno o l'altro?

una proposta di stop assoluto a una diavoleria che aveva inventato il ministro Castelli del centro-destra che si è risolta con una larga sconfitta, diciamolo, dei propositi controriformisti del ministro Mastella. È stato, ancora prima, il decreto Bersani, con cui questo centro-sinistra anche in materia di giustizia è riuscito a litigare con il mondo e a battersi contro il mondo. Oggi abbiamo questo provvedimento che va bene perché tutto

perché trattiamo ancora oggi di una materia che non appartiene né alla destra, né alla sinistra, ma a tutti gli italiani. Sapere allora che tutti gli italiani vedranno regolate le norme che servono a disciplinare le loro ragioni di buona convivenza,

pare, però, che l'idea del decreto-legge in questo caso corrisponda ad una necessità psicologica e pratica. Noi eravamo dinanzi a due fenomeni, uno dei quali cioè quello della pubblicità data a intercettazioni legali, messe però in circolo poi in modo assolutamente arbitrario. Qui rientreremo nel

politico. Noi che apparteniamo al Vecchio Testamento, siamo sempre portati a ricercare dei precedenti. Noi avemmo una stagione nella quale si discusse molto (e vi fu anche una Commissione parlamentare, presieduta dall'onorevole Alessi) sulle cosiddette schedature realizzate dai Servizi e sulle intercettazioni abusive.

stato chiesto dove fossero le prove. Non so se qualcuno di voi ha visto, un paio di settimane fa, la trasmissione «Matrix». Mentana ha interrogato il responsabile di questo servizio di Telecom, il quale ha raccontato tutto.

Tant'è vero che la prudenza dei legislatori è stata tale che, per il sospetto che potesse essere usato in maniera diversa, non è si è dato luogo ad un adempimento previsto dalla Costituzione, cioè la legge sui partiti, perché dalla sinistra si temeva che rappresentasse una specie di schedatura. D'altra parte, si ricordava - vero o no che fosse, forse accentuato che le prefetture giolittiane si impicciavano troppo anche delle elezioni. Quindi non si è mai varata nemmeno quella legislazione, proprio per questa tutela; però a me pare che,

presa di coscienza nei confronti di un'opinione pubblica che è stata turbata. Certamente, è turbata quando si parla di possibili deviazioni dei Servizi, ma

Quando sono venute fuori le intercettazioni, sia quelle paralegali sia quelle abusive, mi è venuto in mente un cartello - qualcuno di voi, se non è giovane, se lo può ricordare - che durante la guerra era esposto in tutti i locali pubblici: «Taci! Il nemico ti ascolta». Mi è tornato in mente, pensando che qualche volta il nemico agisce anche per iniziativa privata.

Signor Presidente, onorevoli senatori, signori del Governo, i fatti, le premesse di fatto, che hanno condotto alla presentazione del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, sono sicuramente e oggettivamente molto gravi. Le cronache giudiziarie, così come riportate e sintetizzate dai *mass media*, danno atto di violazioni pesanti e profonde della legalità democratica. Pur non potendosi in questo momento, per ovvi motivi, dare giudizi su responsabilità personali, è indubitabile che la raccolta illegale di informazioni, notizie, dati concernenti singole persone ha riportato nel Paese un'aria mefitica. Tanto più quanto risulteranno provati l'uso e il ricorso a strumenti di intercettazione e a mezzi tecnologici avanzati. Tanto più quanto sarà confermato il coinvolgimento di esponenti di vertice, di società private e/o di appartenenti ad apparati di sicurezza, ai danni di personalità di rilievo istituzionale anche elevato. Tanto più quanto sarà confermata l'attività illecita e di schedatura spionistica ai danni di tanti lavoratori e anche di semplici cittadini e ciò è in contraddizione con lo spirito e le norme dello Statuto dei lavoratori. Tutti ci siamo sentiti colpiti da questa illecita interferenza nella sfera personale, politica e professionale di singoli cittadini, soprattutto per il fatto che ci sembrava di tornare ai peggiori tempi bui del passato e per il fatto che sono ancora da individuare i cervelli e le finalità precise di tale complessa opera criminale. Bene ha fatto pertanto il Governo a decidere un provvedimento immediato e urgente che, non a caso, ha ottenuto un plauso iniziale pressoché generale. Il fatto però è che, nella materiale e troppo rapida formulazione dell'articolato del decreto-legge che ci riguarda, si sono verificate alcune disfunzioni che hanno generato delle perplessità non solo tecniche e che hanno comportato un lavoro a fondo da parte dei rappresentanti di tutti i Gruppi all' interno della Commissione giustizia. Erano e sono in gioco valori fondamentali per la nostra vita istituzionale e per i nostri rapporti interpersonali: è in gioco innanzitutto la necessità di tutelare la persona, la sua dignità, la sua esigenza di riservatezza, la persona in ogni suo aspetto e in tutte le sue variegate sfaccettature, in ogni sua dimensione. È in gioco la libertà di stampa, colonna portante di ogni democrazia moderna, sono in gioco altri valori costituzionali, come la necessità di svolgere ogni indagine penale fino in fondo e come l'obbligo costituzionale di garantire, all' interno del giusto processo, tutte le parti. Il lavoro compiuto dalla Commissione giustizia, sintetizzato negli emendamenti 1.1000, 2.1000, 3.1000 e 4.1000, ha tenuto ben presente tutte queste esigenze, cercando di contemperare i vari interessi in gioco. In sintesi, questi sono i capisaldi della nuova normativa che dovremmo approvare oggi. Primo: l'immediata distruzione del frutto delle attività criminali che viene disposta da un giudice e non dal pubblico ministero, che in sé rimane parte processuale, così fornendo al cittadino il massimo di garanzia istituzionale. Distruzione che viene disposta in contraddittorio tra le parti, nel corso di un' udienza fissata nell'ambito del presente sistema processuale il più rapidamente possibile; così si vengono a garantire tutte le esigenze, anche processuali, dei singoli cittadini. Secondo aspetto rilevante: dei documenti e degli atti raccolti illegalmente non può essere fatta copia in nessuna forma e in nessuna fase processuale. Terzo aspetto rilevante: il regime giuridico del contenuto degli atti, dei dati, dei documenti raccolti illegalmente è parificato a quello degli scritti anonimi di cui al primo comma dell'articolo 240 del codice di procedura penale. Letteralmente, il loro contenuto non può essere utilizzato come *notitia criminis*, né può assumere valore di prova processuale. Viene peraltro salvaguardata, nel sistema esistente, ed è confermato, la possibilità prevista di trarre spunto investigativo o di prevenzione da tali notizie:

emersa in sede di Commissione affari costituzionali, in riferimento alla fattispecie di cui all'articolo 118 del codice di rito penale. Ulteriore aspetto rilevante è quello considerato dall'articolo 4 del decreto-legge, che prevede la possibilità di chiedere in sede civilistica una riparazione in denaro per tutti coloro cui gli atti e i documenti illegalmente raccolti facciano riferimento, nel caso in cui il contenuto di detti atti sia stato pubblicato. Il meccanismo processuale individuato è stato ispirato alla istituzionale necessità di contemperare gli interessi del cittadino con quelli della libera stampa. Il fatto che sui capisaldi della nuova normativa che vogliamo introdurre si sia trovato un amplissimo accordo è chiaro sintomo, da una parte, dell'estrema sensibilità per una materia così delicata; dall'altra, della consapevolezza generale di dover intervenire con urgenza a regolamentare e a cercare di reprimere gravi comportamenti criminali. Nessuno deve nascondersi e nessuno vuole nascondere il fatto che possibilità di copiare o fotocopiare il materiale illecito, di cui discutiamo, continueranno sempre ad esistere. Sono la nostra storia e la nostra esperienza che ancora una volta ci sono maestre per tutto ciò. Peraltro, questo intervento normativo urgente vuole essere un chiaro segnale di attenzione al problema e all'intera vicenda, nell'intento di porre un argine, per quanto fragile possa essere o rivelarsi; un argine al dilagare di gravi attività criminali che, se non controllate e se non individuate per bene fino in fondo, possono creare rischi e pericoli per la nostra stessa legalità democratica.

Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, ci si è domandati nel dibattito se questo provvedimento sia a tutela del Palazzo o dei cittadini. È del tutto chiaro che noi, come giustamente ha detto la senatrice Boccia, non siamo qui per accertare i fatti, ma per partire da un allarme sociale derivato da fatti che, come ricordava poco fa il presidente Andreotti, sono di pubblico dominio. Da quei fatti emerge che certamente i cittadini comuni, nell'ipotesi di cui si parla, sono stati gravemente colpiti nei loro diritti. Il primo parallelismo rispetto alle vicende del passato, che avremmo voluto non si ripetessero, è la schedatura dei lavoratori della Telecom,

Il secondo triste parallelismo con il passato è il ruolo dei Servizi di sicurezza nella vicenda. Questo punto è molto delicato. delicato. Non dobbiamo accertare i fatti, ma se vi è tutto questo allarme, se si teme un attentato alla democrazia e così via, com'è possibile - lo chiedo al Governo, ma anche a quell'organismo eminentemente *bipartisan* che è il COPACO è il COPACO - che l'allarme sia tale da porre ad un provvedimento d'urgenza profili di costituzionalità, al punto che abbiamo dovuto fare un'operazione di ortopedia per cercare di rimetterlo tutti insieme nei binari della legge,

terza osservazione che è stata avanzata è che non si parla delle intercettazioni. Il Governo ha presentato un altro disegno di legge, a suo tempo, e ha ritenuto, nella sua saggezza, di portarlo nell'altro ramo del Parlamento, dove non mi risulta sia iniziato l'esame; l'esame; il bicameralismo comporta che noi ci si debba occupare di quest'altra materia (non che l'altra non abbia un suo peso ed un suo rilievo). Infine, onorevoli colleghi,

la lettura del testo potrà rassicurarlo, perché entrambe le questioni da lui sollevate - cioè la genericità del termine «divulgazione» e l'entità, ritenuta eccessiva, della pena pecuniaria - sono state oggetto dell'intervento emendativo della Commissione.

su questo tipo di questioni non si intervenga solo sull'onda dell'emozione e dei titoli, dei quotidiani, ma vi sia trasparenza, vi sia un'attenzione continua perché vi sia trasparenza nella vita pubblica e perché la garanzia della tutela della riservatezza dei cittadini, a cominciare da a cominciare da quelli comuni, sia protetta e lo si faccia, com'è possibile farlo - e come abbiamo cercato di fare con i nostri emendamenti - senza mettere in discussione princìpi basilari del nostro ordinamento democratico come il giusto processo, il diritto alla difesa, l'obbligatorietà dell'azione penale. A mio avviso, il testo condiviso in Commissione consente di tutelare l'esigenza per far fronte alla quale il Governo ha ritenuto di proporre la decretazione di urgenza, salvaguardando, al tempo stesso, il rispetto dei princìpi costituzionali. Credo quindi che consegniamo al Senato un testo

Signor Presidente, signori senatori, le ragioni che hanno indotto il Governo a presentare il decreto‑legge sono state ripetute abbondantemente in quest'Aula e quindi non posso che non posso che riportarmi a ciò che è stato già detto. Peraltro, quella del Governo era una decisione ampiamente condivisa da tutte le forze politiche, appositamente consultate, tant'è che le prime reazioni

positive. Forse qualche errore nel dibattito si riesce a cogliere nel momento in cui si accentra il discorso sul tema delle intercettazioni illegali.

quella delle intercettazioni telefoniche illegali. Sappiamo benissimo che sia le intercettazioni illegali, sia le intrusioni nella vita privata, sia la violazione della corrispondenza sono già tre profili di reità codificati ed esistenti nel Codice. Quello che il Governo ha ritenuto di dovere fare è coprire quella zona d'ombra non sanzionata e non prevista dal legislatore, ossia il provento di queste condotte illecite, attuate attraverso le intercettazioni, la captazione abusiva nella vita privata e anche la violazione di corrispondenza, senatore Palma, nel senso che si riferisce a tutte quelle condotte che consentono all'autore dell'illecito di produrre poi qualche cosa di altro che potrebbe portare alla commissione di ulteriori condotte.

forma riparatoria e risarcitoria in favore delle parti interessate. È stato posto il problema il senatore Castelli ne ha fatto oggetto dei quattro paradossi, attribuiti al Governo.

proceduto ad emendare il suo testo. In verità, la decisione del Governo era di affidarsi al lavoro della Commissione,

che prevedeva la possibilità della distruzione differita a diciotto mesi o, addirittura, della non distruzione, perché necessaria al rispetto del principio della formazione della prova nel dibattimento

che almeno, qualora si fosse differita la distruzione di tale materiale illecitamente formato, prevedessero comunque la possibilità di alcuni presidi normativi a tutela dei terzi (e cioè che, nel momento in cui tale materiale veniva travasato in un procedimento penale, esistessero comunque alcuni presìdi). La presentazione degli emendamenti - com'è noto - ha provocato giustamente, legittimamente e comprensibilmente richieste di approfondimento da parte dei componenti delle Commissioni affari costituzionali e giustizia, il che avrebbe potuto determinare uno scivolamento dei lavori programmati di quest'Aula. Per tale ragione, il Governo ha deciso

Ovviamente, il risultato cui è pervenuta la Commissione è per noi soddisfacente: volevamo prevedere una nuova fattispecie di reato, ed il punto è stato mantenuto fermo; volevamo prevedere la distruzione del materiale illecitamente formato, e tale previsione è stata recepita dalla Commissione; volevamo prevedere una forma risarcitoria e riparatoria per la parte interessata che avesse subito danni da tali iniziative illegali. In questo senso, quello svolto dalla Commissione

una tutela delle intercettazioni illecite delle comunicazioni o dei flussi telematici, ma non della conoscenza illecita della corrispondenza privata.

con il presidente Salvi quando egli contesta l'affermazione, che ho cercato di motivare in discussione generale, che questo decreto-legge sia un provvedimento destinato

alla Camera. Il collega Salvi ha voluto cercare di mitigare la mia affermazione un po' radicale, sostenendo che questo provvedimento riguarda anche la schedatura dei dipendenti Telecom. Dobbiamo non essere ipocriti e riconoscere

per rendere possibile l'immediata distruzione di ciò che è stato illegalmente acquisito, si manda fuori dallo squadro complessivo

mera riproduzione in un apposito verbale, che non può assolutamente riguardare il contenuto degli atti, possa essere un surrogato che consenta di sviluppare le indagini, di garantire la parte lesa, di assicurare che l'esercizio obbligatorio

rispondere, quanto meno in concorso, con colui il quale detiene, in qualche modo, il materiale, la facciano franca. È un prezzo che si paga. Vorrei che tutti fossimo consapevoli di questo prezzo che viene chiesto alla nostra democrazia. In questa logica, Presidente, è stato presentato il mio emendamento abrogativo.

e non capisco questa regressione intempestiva che si ha in Aula a quale disegno soggiaccia. Avevamo convenuto sull'introduzione dell'avverbio «consapevolmente» perché riteniamo che in questa fattispecie, che è fattispecie autonoma, l'inserimento dell'«illecitamente» serva esclusivamente a connotare di una particolare intensità il dolo richiesto dalla norma e quindi praticamente serve a rendere non punibili gli autori di questo illecito.

Si era arrivati alla necessità di verificare il momento dichiarativo di questa illiceità, che ovviamente non può essere che il provvedimento di distruzione del GIP che accerta questo tipo di illiceità. Cosa succede nel momento precedente all'emissione di questo provvedimento, cioè per chi ha detenuto documenti che fino ad allora comunque non sono classificabili, ai sensi di legge, come illeciti o illegittimi, perché lo stesso GIP può sempre verificare la liceità dei documenti sequestrati ad una persona? Evidentemente vi è una sorta di retroattività della dichiarazione che copre il momento antecedente per il quale vale l'avverbio della illiceità, mentre per il periodo successivo vi è comunque il provvedimento che fa stato sulla illegittimità. Queste sono le ragioni di questa modifica che certamente ha ampliato lo spettro e ha coperto anche una zona che era rimasta scoperta perché, diversamente, chi, nel periodo precedente al provvedimento di distruzione, comunque aveva questi questi atti, queste intercettazioni illecite, non era passibile di alcuna pena perché non vi era un provvedimento che ne sancisse l'illegittimità: era un momento di assoluta impunibilità e quindi da qui la necessità di questa ulteriore aggiunta fatta in corso d'opera, in Aula.

una volta che viene dichiarato il sequestro e che è stato detenuto prima del sequestro, costituisce sostanzialmente reato mi sembra, sotto il profilo dei princìpi generali, una stranezza. Una cosa è parlare di chiunque detiene chiunque detiene documenti di cui è stato ordinato il sequestro: *nulla* *quaestio*, ma dire «ha detenuto» è un problema anche perché, Presidente, forse ci si dimentica

Mi permetto di farle rilevare, senatore Palma, che la questione dirimente non riguarda il tempo della detenzione, ma l'«illecitamente» ovvero il «consapevolmente». Mi pare che questo sia il punto sotto il profilo non politico ma giuridico-formale più rilevante.

punibilità di chiunque detenga atti o supporti per i quali è disposta la distruzione ai sensi dell'articolo 240 del codice di

e magari inviata a tutti, determina la mera detenzione. Come facciamo noi a comprendere se quella determinazione rientra nella previsione criminale che con questo articolo viene fatta? Dovremmo sapere se

la mera detenzione configura un'ipotesi di reato oppure no? Vorrei che questo ci venisse spiegato. Siamo ancora all'interno del solco dell'originario decreto-legge fatto, e lo ribadisco, per coprire i piani alti di alcuni palazzi rispetto ad un abuso abnorme, quello della Telecom, comportante una serie di abnormità che poi sconteremo. Stiamo introducendo nel nostro sistema giuridico un regime differenziato che non guarda alle regole ordinarie e cerca di inserirsi all'interno di un tessuto connettivo giuridico già collaudato, ma che pone priorità diverse, in questo caso quella di punire e scoraggiare la mera detenzione, prevedendo delle aberrazioni che ci verranno contestate.

una riformulazione che tiene conto, fra l'altro, dei rilievi mossi dalla Commissione affari costituzionali nell'intervento del senatore Villone. Segnalo che la sanzione è prevista nell'ipotesi di pubblicazione e non di mera divulgazione come, invece, previsto nel testo originario - e che la pena minima è stata dimezzata rispetto alla previsione originaria del decreto-legge, onde evitare, soprattutto per i giornali minori, locali, o per radio locali, che la sanzione pecuniaria potesse essere di entità sproporzionata al danno arrecato.

che vorrei illustrare. Pregherei soprattutto i colleghi della Casa delle Libertà di fare un ultimo sforzo per ascoltarmi, perché credo che il tema non sia secondario. Cosa stiamo facendo oggi? Nella *vulgata*, come viene riferito dai *media*, il cittadino comune è convinto che stiamo intervenendo per sanare quel problema che viene definito, con termine popolare, lo scandalo delle intercettazioni telefoniche, cioè quello scandalo per il quale vengono propalate, lette sui giornali e viste in televisione intercettazioni telefoniche che riguardano soggetti che nulla hanno a che vedere con l'inchiesta, che entrano nella vita privata delle persone, che alcune volte hanno rovinato persino delle vite. Non stiamo facendo questo, colleghi, questo è molto importante. Non lo stiamo facendo perché tutti i casi di cui ci siamo occupati in questi anni riguardano intercettazioni telefoniche legalmente e legittimamente acquisite acquisite su ordinanza dell'autorità giudiziaria. L'illecito avviene dopo, nella loro propalazione. In questo caso non affrontiamo questo tema, ma ci occupiamo, come prevede

al traffico telefonico o telematico illegalmente formati o acquisiti. Ci occupiamo quindi di tutt'altro: si tratta di casi meramente virtuali perché fino a questo momento non si ha notizia che ciò sia accaduto

di vecchie lire dei cittadini - questo il costo di tale seduta - facendo finta di lavorare e facendo credere ai cittadini che interveniamo su questo scandalo che abbiamo visto sui giornali in tutti questi anni. Non è però

di casi che al momento non esistono o di cui, se esistono, non siamo a conoscenza, a meno che non ne sia a conoscenza il presidente Prodi o qualche Ministro, data la fretta assoluta con cui sono intervenuti. C'è anche da domandarsi come mai il presidente della Repubblica Napolitano abbia firmato un decreto di cui non si capisce l'urgenza. Non so se è chiaro il tema di cui stiamo trattando. trattando. Gli emendamenti che ho proposto non sono altro che gli articoli del testo di legge approvato dal Governo Berlusconi nel settembre 2005 trasformati in emendamenti.

tratta, quindi, una questione molto importante. È strano che la Commissione giustizia del Senato abbia avviato un'indagine conoscitiva sulla materia e poi il Ministro abbia fatto approvare dal Consiglio dei ministri il testo di un disegno di legge su questo tema, di cui parlano i miei emendamenti, e lo abbia presentato alla Camera. Credo che forse per un po' di correttezza istituzionale, Ministro, valeva la pena che lo presentasse al Senato. Questo è il dato, altrimenti altrimenti abbiamo l'impressione di lavorare per nulla a meno che non intendiamo poi, avendo acquisito una serie di conoscenze, ribaltare il testo che

innanzitutto di ringraziare il senatore Valentino del mio Gruppo per averla anticipata. Vorrei spiegare la motivazione di questo emendamento, su cui poi chiederò una votazione elettronica,

Presidente Angius, coincidenza vuole che questa seduta sia presieduta proprio da lei. Il mio è stato un calvario personale iniziato un giorno che eravamo in diretta televisiva. Vorrei indicare con molta chiarezza all'Assemblea - se mi si consente di parlare - alcune questioni. Ho trattato questo problema ad una festa di partito, quella dell'Italia dei Valori. Annunciai la presentazione di un disegno di legge, mai discusso in Commissione giustizia, sulla sottrazione dei membri del Parlamento ai benefici dell'indulto. Questo disegno di legge, senatore Salvi - spero che prima o poi la Commissione abbia il tempo e il modo di esaminarlo serve a far capire proprio quello che lei ha poc'anzi affermato. I parlamentari godono già di privilegi rispetto ai cittadini: sarebbe sbagliato sommare privilegi a benefici, o almeno questa è la mia opinione personale. Oggi discutiamo sul tema delle intercettazioni. Sette mesi fa, a seguito di una vicenda montata - come dimostrano gli atti giudiziari, finalmente depositati - mi sono dovuto dimettere da ministro. Rivendico con orgoglio quella scelta, perché non bisogna mai ostacolare il lavoro della magistratura.

Abbiamo letto sui giornali di altri illustri esponenti politici, come il segretario dell'UDC, onorevole Cesa, e l'onorevole Mirko Tremaglia, che figurano tra gli elenchi dei pedinati. pedinati. Non so quanto sia grave lo spionaggio industriale ed è sicuramente grave lo spionaggio ai danni dei dipendenti; ma, signor Presidente, credo che lo spionaggio politico sia una questione di democrazia, sia pericoloso per la democrazia.

Se dovesse punire chi ha commissionato intercettazioni e se quelle intercettazioni fossero state commissionate da esponenti politici, la farebbero franca o no, visto che l'indulto non ha escluso questa fattispecie di reato? reato? Colleghi, discutiamo di una cosa importante. Lo dico anche perché sono rimasto ferito personalmente da notizie diffuse dalla procura della Repubblica di Roma. Si diceva che l'indulto salvasse anche vicende accadute all'epoca in cui mi sono dimesso da Ministro e non era vero, perché sono scomparsi i capi di imputazione. però, che ci sia qualcuno che può essere ancora imputato per aver spiato avversari politici: l'indulto lo salverebbe. Ecco perché ho presentato questo emendamento, che serve ad escludere i membri del Parlamento dai benefici della legislazione dell'indulto, proprio per quello che diceva il presidente Salvi poc'anzi: non diamo l'impressione del Palazzo che si difende. Ecco perché è importante dedicare

anche perché non possiamo lasciare che spiri il venticello della calunnia. Vi è stato un giornale che ci aveva provato: «la Repubblica». Questo giornale non lo farà più. Credo che il Parlamento debba poter difendere l'onorabilità di ciascuno dei membri dell'Assemblea.

Il Governo è sovrano nel decidere a quale dei due rami del Parlamento inviare la materia: se lo ha inviato alla Camera dei deputati avrà avuto le sue buone ragioni che non conosciamo, ma sicuramente nella sua saggezza il Ministro avrà ritenuto di far bene, dunque non possiamo cambiare questa situazione.

nel quale si è introdotta la figura della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e anche di altri enti e associazioni che non siano persone giuridiche, ma abbiano condizioni assimilabili. La valutazione è stata questa: molto spesso di fronte a fattispecie che, se commesse da una persona fisica avrebbero comportato le pene tradizionalmente previste, non si è in grado di intervenire, perché in realtà il "reato" è stato commesso da una persona giuridica.

ci fossero fattispecie a proposito delle quali fosse giusto prevedere la responsabilità di un ente e non solo di una persona - ipotesi delittuose,

Però questa è una norma di cui sempre si è detto che l'entità minima della sanzione prevista comporti sostanzialmente l'irrilevanza della norma stessa. Essa si riferisce a chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, alla cosa che accade quotidianamente e di cui si dice non ci siano strumenti per contrastarla. In realtà, essa è prevista come reato, ma essendo la pena o l'arresto fino a 30 giorni o l'ammenda sino a 258 euro, si tratta di una sanzione che praticamente non ha caratteristiche deterrenti. Se aggravarla o meno rispetto alla persona fisica è una questione delicata, perché c'è la libertà di stampa. Il senatore Castelli propone di applicare in questa ipotesi la responsabilità amministrativa dell'ente: si

che sono già previste come contravvenzione ma con una pena minima - si applichi una sanzione pecuniaria come già previsto nel sistema. Si parla

potrebbe prevedere una sanzione pecuniaria fino a 150, per la stessa ragione per cui abbiamo rivisto la norma sul punto. Mi rimetto al Governo innanzitutto che può dare una valutazione su questo e poi all' Assemblea come relatore.

questa legge in realtà, come nuovo reato, prevede soltanto la detenzione illecita, di cui sopra, naturalmente dal momento in cui entra in vigore. Tutto quello che è accaduto in precedenza, per l'ovvio principio della successione delle leggi penali nel tempo,

Per quanto riguarda l'emendamento 4.0.2, faccio presente che viene introdotta una disciplina l'articolo 25-*septies* che riguarda, subito dopo, il reato di abusi di mercato. Non solo; si prevede il riferimento all'articolo 684 del codice penale che riguarda la pubblicazione di atti di un procedimento penale. Penso che vi sia francamente un bisticcio tra la norma che si intende inserire penale che riguarda la pubblicazione di atti di un procedimento. Non solo. Ritengo la norma particolarmente pericolosa perché, qualora dovesse spostarsi questa sanzione sull'editore, potremmo avere quale conseguenza l'interesse dell'editore a preventivamente censurare l'esercizio della libertà di informazione del giornalista al fine di evitare il rischio. Quindi, potremmo inserire un qualcosa di esattamente contrario

ovviamente una tipologia di reato, sia perché ritengo la norma inserita in questo contesto del tutto sproporzionata rispetto alle sanzioni già previste all'articolo 4 del decreto-legge in esame.

Scusi, signor Sottosegretario, questa è una sua autorevolissima opinione, ma non corrisponde all'opinione della Presidenza del Senato. Infatti, la Presidenza del Senato dichiara ammissibile l'emendamento perché, mentre l'articolo 79 della Costituzione fa riferimento ad un regime concessorio dell'indulto, qui siamo in un regime di limitazione dell'indulto medesimo.

è l'ultimo intervento che faccio di questa rappresentazione de «Il Palazzo si tutela»; siamo arrivati a «Il Palazzo si tutela 4». Abbiamo visto che il Palazzo si tutela prevedendo un regime giuridico diverso da quello ordinario; abbiamo visto che si inventa un reato aggravato, come la mera detenzione, rispetto alla figura ordinaria che viene trattata diversamente, dove è prevista una perseguibilità a querela. Adesso il Palazzo si tutela rispetto alla possibilità di ottenere la riparazione del danno, o meglio il risarcimento. Non comprendo perché una norma come questa, che velocizza la possibilità di ottenere il ristoro dal danno subìto con la pubblicazione, non sia una norma che venga immaginata a regime per tutti i casi di diffamazione a mezzo stampa. Se questa fosse stata la proposta del Governo, non avrei avuto nessuna difficoltà a condividerla. Quando una proposta come questa nasce soltanto («Il Palazzo si difende 4», dicevo poco fa) per coloro i quali siano stati colpiti dalle intercettazioni illegali, che sappiamo quali figure tocchino (l'ho detto all'inizio della discussione) e non tutti gli utenti della giustizia, allora mi chiedo perché dobbiamo immaginare questo circuito particolare che prevede una serie di accelerazioni, secondo me ingiustificabili. Infatti, se si trova un percorso che determina l'accelerazione nella soluzione di una pretesa, nel fare in modo che un diritto venga tutelato, allora questa accelerazione deve valere per tutti. Se vale solo per alcuni, rimane il sospetto che si voglia creare una corsia privilegiata. Vedete, la stessa confusione con la quale si sta andando avanti, Presidente (non è un appunto alla Presidenza; mi riferisco al fatto che molto spesso si propongono riformulazioni che poi, in effetti, sono modifiche emendative significative che poi si ritrattano), dà l'impressione di come purtroppo lo strumento del decreto‑legge non sia stato uno strumento adeguato rispetto ad una normativa che sicuramente avrebbe meritato un approfondimento diverso. Se la logica, però, è sempre la stessa, tutelare il Palazzo, mentre prima si cercava di colpire la detenzione, adesso si cerca di scoraggiare i giornalisti con una normativa che, proprio perché accelerata, favorisce il diritto ma ha una forza di intimidazione nei confronti della stampa molto maggiore. in tale logica, continuo a chiedermi se esistano le condizioni generali per ritenere che alcuni siano cittadini di serie A (quelli del Palazzo e dei piani alti)

ringrazio la Presidenza del Senato per aver chiarito la questione legata all'ammissibilità dell'emendamento. Non ho la competenza giuridica del presidente Salvi, al quale chiedo un attimo di attenzione. Vede, presidente Salvi, uno dei dubbi che ho sul decreto‑legge in esame riguarda proprio la natura del reato che si commette: si dice che da oggi si viene puniti perché si commette questo nuovo reato (come vede, parlo in termini molto semplici, come un cittadino comune). Voglio immaginare che, nel momento in cui vengano trovate in casa di un cittadino comune intercettazioni ad un tizio, tale cittadino venga perseguito, le intercettazioni vengano distrutte e qualcuno gli chieda chi gliele ha commissionate.

intervengo per dichiarare che sosterremo l'emendamento presentato dal senatore Storace, non foss'altro perché crediamo che rientri in un'ipotesi che formulammo all'epoca del voto sull'indulto, al quale ci opponemmo con tutte le nostre forze parlamentari.

capimmo che probabilmente esso avrebbe avuto anche una valenza a futura memoria e volevamo evitare che ciò potesse avvenire. Ci opponemmo anche - se non soprattutto - per questo motivo. Credo che l'ipotesi tracciata all'Aula

dubito che possa avere una qualche efficacia, ma questo poi lo si vedrà. Vorrei, però, invitare il senatore Storace, depositario e proponente dell'emendamento,

e tutti i pubblici ufficiali abbiano una responsabilità di natura etica, quindi anche giuridica, pari ai membri del Parlamento. Io voterò l'emendamento in ogni caso, ma lo voterei più convintamente se il senatore Storace volesse accogliere questa riformulazione.

pregevole negli intenti, è tecnicamente inapplicabile per il semplice motivo che recita testualmente che: «Le violazioni alla presente legge

fa sì che vi sia la punibilità soltanto nei casi in cui si detengano «consapevolmente» dei documenti di cui sia stata disposta la distruzione. È evidente, dunque, che non v'è nessuna forma di reato per la detenzione pregressa alla disposizione che questa documentazione venga distrutta (ciò che il subemendamento proposto dal presidente Salvi voleva evitare). È evidente quindi che non vi può, in alcun modo, essere un'applicazione dell'indulto, dell'indulto, perché l'indulto si ferma soltanto ai reati commessi antecedentemente alla data fissata dal Parlamento.

a me sembra chiaro, cari colleghi, che le violazioni alla legge che noi ci accingiamo a varare ora in Parlamento presuppongono l'entrata in vigore di questa legge, sono ad essa successive. Non si capisce, quindi, come a queste violazioni possa applicarsi la norma sull'indulto che riguardava i fatti anteriori al 4 maggio 2006.

accertare con chiarezza le responsabilità per fatti di spionaggio politico, per raccolta illecita di informazioni in un'epoca anteriore anteriore alla norma sull'indulto (e credo che egli a quello faccia riferimento perché la vicenda che noi conosciamo, che riguarda il Lazio, implica una collaborazione tra

rispetto alla quale ci siamo divisi (l'orientamento del collega Storace e di altri colleghi era infatti contrario). Noi abbiamo detto che con l'indulto non si cancella nulla ed è su questo punto che vorrei insistere. In particolare, se si accerterà che vi sono dei politici responsabili di attività spionistiche, in tutte le direzioni possibili, vi sarà l'accertamento delle responsabilità, come vi sarà la riprovazione, dentro e fuori del Parlamento. questo possa bastare, non facciamo il tifo per la galera. Certo, se ci fosse stata l'amnistia, sarebbe stato diverso, ma riteniamo che l'indulto non cancelli nulla e quindi, anche per quei fatti che non c'entrano con quelli di cui stiamo discutendo, anche per quella vicenda è giusto esigere che si accertino tutte le responsabilità,

Rispettosamente, chiediamo alla magistratura competente di rassicurare quanto prima i cittadini e le istituzioni in ordine a quella vicenda che riguardava il Lazio, e cioè la Regione di cui è stato

del senatore Storace abbia raggiunto l'obiettivo, quello cioè di sottolineare per l'ennesima volta il danno che è stato provocato dal provvedimento sull'indulto che il Parlamento ha varato qualche mese fa; però che, al di là di questo effetto, non ne possa produrre altri. Non valgono infatti soltanto le considerazioni tecniche che sono state svolte dal senatore Ghedini e, se ho ascoltato bene, anche dal senatore Brutti, ma anche una considerazione elementare che chiama in causa la successione delle leggi penali nel tempo e quindi gli articoli 2 del codice penale e 25 della Costituzione. Purtroppo - dico purtroppo perché l'ho osteggiato - l'indulto ha avuto operatività e questa è una normativa più favorevole non soltanto rispetto alle condotte che saranno poste in essere in violazione di tale legge, che sono automaticamente escluse per via del *dies a quo* dell'entrata in vigore dell'indulto, ma anche per quelle antecedenti che cadono sotto altre norme incriminatrici, qualora rientrino nelle disposizioni coperte dall'indulto. Peraltro, Parlamento può fare tutto, ci mancherebbe altro, ma normalmente in una disposizione generale sull'indulto si possono inserire delle eccezioni; sarebbe forse la prima volta

la discussione ha fatto emergere la circostanza che probabilmente fatti molto gravi che chiamano in causa spionaggio industriale e politico saranno coperti dal provvedimento di indulto.

«il Presidente può stabilire, con decisione inappellabile, la inammissibilità di emendamenti privi di ogni reale portata modificativa». Ora, se mettiamo in votazione l'emendamento, ciò significa che esso ha portata modificativa, e quindi la richiesta avanzata dai senatori Ghedini e Brutti al senatore Storace non ha ragion d'essere. Se invece la Presidenza non lo mette in votazione, ciò significa che hanno ragione i senatori Brutti e Ghedini. Pertanto, indipendentemente dal dibattito che c'è stato, se la Presidenza decidesse in tal senso si eviterebbe di dover mettere in votazione la Presidenza non può entrare nel merito di considerazioni di carattere politico e di opportunità. Nel momento in cui si è dichiarata l'ammissibilità dell'emendamento medesimo e nel momento in cui

Fatemi dire, cari colleghi, che la discussione che c'è stata - e voglio ringraziare il senatore Storace e tutti coloro che sono intervenuti - ha fatto dare al Senato una piccola prova di civiltà politica, alla quale non sempre siamo abituati. Vorrei ringraziare pertanto tutti i colleghi.

quindi si presume che, una volta che il Presidente, o chi per esso, abbia effettuato la sua dichiarazione a nome del Gruppo, poi il Gruppo voti di conseguenza. Ora, l'Italia dei Valori ha votato in maniera difforme dalla dichiarazione del Capogruppo perché ho notato che soltanto un voto è stato a favore, quando l'Italia dei Valori ha dichiarato che avrebbe votato a favore.

Vengo al tema in questione. Io ringrazio il relatore per avere, se non accolto, comunque esaminato con grande attenzione e non con sfavore questa fattispecie. Vorrei invece interloquire con il sottosegretario Li Gotti che si è dichiarato contrario. A

delle vicende assolutamente private e personali, desunte da intercettazioni illegalmente propalate che nulla hanno a che vedere con le vicende giudiziarie e servono semplicemente a squalificare dei privati cittadini.

incinta e di due signori che facevano apprezzamenti di natura sessuale su questa signora riportati nel 1996 dal più grande quotidiano italiano. Bene: per questa cosa il quotidiano oggi oggi pagherebbe 50 euro, allora pagava 100.000 lire di sanzione. Io credo che questo non sia assolutamente giusto. A cosa mira la nostra proposta? Intanto credo che sia estremamente moderna

Spesso queste notizie vengono pubblicate soltanto per soddisfare la sete di *gossip* dei lettori, che esiste. Quindi, ne trae vantaggio ne trae vantaggio il giornalista, perché si fa bello presso l'editore, ma soprattutto ne trae vantaggio l'editore stesso, che aumenta la tiratura della propria edizione e non paga nulla. Con questo sistema si introduce una sanzione che è a discrezione del giudice.

per quel giornale che non esercita più la libertà di stampa ma l'arbitrio, la violenza sulla *privacy*, delle persone, oggi con totale immunità.

società e gli enti a vario titolo in corrispondenza ad una serie di reati che, nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, vanno dalla concussione e corruzione, alla falsità in monete, ai reati societari, ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ai delitti contro la personalità individuale, agli abusi di mercato. Si è, cioè, ipotizzato che, per tutto questo spettro complessivo di reati della più varia fattispecie, vi possa essere anche una responsabilità amministrativa per l'ente che esprime colui che è stato l'autore di questo reato.

dei quali sia ordinata la distruzione è chiaramente vietata per legge: sono comunque atti di un procedimento e tutto avviene nell'ambito di una società, di un'impresa, di un ente. Non c'è alcuna compressione del diritto di informazione, perché siamo comunque di fronte ad un reato

legislativo n. 231 del 2001 è l'unico tentativo moderno e avanzato del nostro sistema per evitare e prevenire la commissione dei reati piuttosto che ricorrere alla sanzione come unico strumento di regolazione della legge. si fonda non su una responsabilità oggettiva dei titolari dell'impresa, dell'amministratore delegato piuttosto che del Presidente o dei componenti del consiglio di amministrazione, perché la responsabilità oggettiva, sia pure in forme limitate ma specificamente nel campo dei delitti riguardanti l'informazione, è già prevista nel codice penale del 1930; il decreto legislativo n. 231 imputa una responsabilità amministrativa alle imprese in forma pecuniaria ogni qualvolta i gruppi dirigenti di tali imprese o enti non abbiano posto in essere un sistema organizzativo e di controllo in grado di prevenire comportamenti commessi da loro dipendenti. Questo sistema, Questo sistema, come voi sapete proveniente da un'elaborazione di livello europeo, è stato previsto originariamente per prevenire ed enfatizzare la responsabilità, la capacità di controllo e la cura nel controllo, da parte

Castelli, troverei utilissimo, nel lavoro che si sta facendo alla Camera, prevedere un tipo di responsabilità di questo genere per la prevenzione di tutti i reati che riguardano, per esempio, l'effettuazione di intercettazioni illegali da parte di imprese che esercitano un'attività

per la ragione che agirebbe ancora una volta - e capisco che questo è l'intento - come una forma di responsabilità oggettiva da parte dell'editore che già esiste, non solo nelle forme in cui è prevista dal codice penale, ma anche perché nello stesso emendamento della Commissione è prevista una responsabilità dell'editore e, quindi, un obbligo al risarcimento del danno della parte offesa secondo le modalità che, d'accordo, si sono stabilite in Commissione. Pertanto, pur trovando molto interessante il fatto che sia stata sollevata da lei, presidente Castelli, la possibilità di utilizzare questo strumento,

Ritengo, peraltro, che la materia sia sufficientemente e aspramente già coperta sia dalla previsione del codice penale sia dalla previsione che introduciamo adesso. Per questo, i senatori del Gruppo

Prendo atto che quel tentativo è andato a vuoto e che siamo in un bicameralismo perfetto per cui questo ramo del Parlamento ha tutta la facoltà,

indiscriminato delle conversazioni telefoniche. Con la riorganizzazione della normativa si pone fine all'Italia degli spioni e degli spiati, riconducendo nei ranghi della legalità tutte le informazioni in qualsiasi modo raccolte, a prescindere dalla premeditazione dolosa o dalla mera casualità. Con ciò non voglio affermare che la giustizia non possa adeguatamente servirsi dei moderni mezzi d'indagine, né però che possiamo accettare il machiavellico «fine che giustifica i mezzi». Vorrei con estrema pacatezza analizzare l'insieme dei punti. Il decreto, infatti, interviene sulla disciplina codicistica dell'acquisizione delle prove, ribadendo il limite dell'utilizzo di quelle ottenute illecitamente ed introducendo quel *quid pluris* che rende necessaria e dovuta la sua conversione. Mi riferisco in particolare all'articolo 240 del codice di procedura penale, risultante dagli incessanti lavori di queste ore, che mantiene inalterati gli elementari princìpi di libertà giuridica anche nel rispetto di altre norme penali. Si introduce la novella che impone l'immediata custodia dei fascicoli illegalmente formati o acquisiti, vietandone, comunque, le copie e rendendone inutilizzabile il contenuto. Questa novella si inserisce in un quadro sistematico teso al totale rispetto della normativa n. 196 sulla *privacy*, anche perché al pubblico ministero, di concerto con il GIP, è lasciato il compito di decidere l'eventuale efficacia probatoria delle intercettazioni e dei tabulati telefonici esistenti. A mio parere questa legge sottende un *modus* *operandi* assennato, che nasce dall'esigenza di rispettare la gerarchia dei valori a tutela dei diritti soggettivi e della persona. Pertanto, anche sotto il profilo della costituzionalità, sostengo che si è rispettato l'articolo 111 della Costituzione, che impone che l'acquisizione della prova avvenga in contraddittorio tra le parti. Inoltre, l'articolo 3 del decreto, dovuto corollario della riforma, prevede una nuova ipotesi di reato, con pena detentiva nel caso di illecita detenzione degli atti e dei documenti. Basterebbe non aggiungere altro, perché appare logico procedere alla conversione di tale decreto, che pone un serio caposaldo nei poteri di indagine e di inchiesta. Tuttavia, a fronte delle preoccupazioni dell'ultimo momento e avendo mediato con le altre forze politiche per addivenire a un miglioramento e ad un consenso vasto, abbiamo accolto le modifiche - come dicevo - migliorative, per rendere più organico il provvedimento che stiamo per votare. Così concludo. Mi sembra che obiettivo primario del decreto legge sia garantire tutti i cittadini, dando loro la dovuta serenità. Pertanto, le finalità che hanno spinto il Governo ad emanare un simile provvedimento d'urgenza sono evidenti e da ricercare nell'inevitabile *stop* alla prassi delle pubblicazioni indebite. Ecco perché, a nome del Gruppo Misto-Popolari-Udeur

riscontriamo un consenso importante su un provvedimento in materia di giustizia. Forse non era prevedibile che in questo ramo del Parlamento, proprio attorno a un tema così delicato, si sviluppasse un dialogo politico che sta producendo risultati apprezzabili. L'utilizzo dello strumento del decreto‑legge da parte del Governo non ha favorito

e di urgenza, visto il vasto allarme sociale che si è determinato in questi mesi attorno al tema delle intercettazioni e dell'acquisizione in forma illegale di questo livello di informazioni. Credo che dalla preoccupazione per una violazione diffusa della *privacy* dei cittadini - per quanto ciò devasti lo spazio personale e individuale con gravi danni - ma probabilmente anche che è stato colto un pericolo più grave, quasi di inquinamento della vita democratica. Alcune vicende palesate in questi mesi hanno forse costituito l'occasione per una riflessione comune

riportato alla memoria antiche vicende che costituiscono pezzi oscuri della nostra storia civile. Ebbene, talmente grave è stata questa preoccupazione, talmente diffusa la volontà di far prevalere queste esigenze e la tutela dei diritti costituzionalmente garantiti, che in sede di Commissione si è sviluppato un percorso che ha fatto prevalere questo, rispetto, ad esempio, sulla possibilità di utilizzare gli esiti di tali attività per accertare eventualmente dei reati. Voglio ricordare che nel dibattito politico, qualche mese fa era apparsa la proposta di utilizzare comunque questi reperti per individuare ed accertare reati. Forse ciò era il frutto ultimo, da parte di qualche esponente di una subcultura inquisitoria, della volontà di ribadire un clima che ha segnato questo Paese.

mettendoli a disposizione dell'autorità giudiziaria. Al contrario, con un clima assolutamente *bipartisan* che si era già

certamente più importante, dell'utilizzo illegale delle intercettazioni acquisite legalmente all' interno dei procedimenti penali, che rappresenta il vero tema che ha visto in questi anni segnare spesso un confronto aspro tra la politica e la magistratura e un utilizzo dei *mass media* qualche volta spregiudicato. Il tema comunque è ormai alla portata del dibattito parlamentare, infatti avviato alla Camera dei deputati: probabilmente, per l'attività che era stata svolta in questo ramo del Parlamento e per il clima che qui si era innestato, forse sarebbe stata anche più giusta un' omogeneità

sul terreno della giustizia sia stato segnato forse il momento di maggiore criticità della storia politica di questi ultimi anni del nostro Paese; che vi sia la necessità da parte di tutti di uno sforzo in avanti, fuori da schematismi ideologici e, sopratutto, da scontri faziosi e partigiani. È necessario rintracciare un filo comune. Il nostro piccolo Gruppo parlamentare, che mette insieme culture diverse e che forse è una sorta di piccolo laboratorio del confronto e della dialettica politica (democristiani, repubblicani, autonomisti; espressione quindi di formazioni e di culture diverse, ma che sono tutte incentrate nel segno della garanzia e della profonda legalità), collaborerà per instaurare questo clima, non soltanto votando convintamente il provvedimento, ma confermando e rafforzando questo spirito. Su tutte le tematiche di respiro istituzionale, ma soprattutto sulla giustizia, i provvedimenti devono essere accompagnati dal più largo consenso che non è soltanto a garanzia di contenuti condivisi, ma è anche piena e assoluta garanzia di una cultura democratica che in questo nostro Paese ogni tanto è stata tanto è stata offuscata e che, invece, va riportata integralmente nel dibattito politico.

prima. Probabilmente, abbiamo avuto momenti di dibattito, non dico alto ma comunque fuori del normale e dell'usuale. Se ci abituiamo a discutere in questo modo, facciamo cosa giusta e saggia per il compito che il Senato ha davanti. Credo di dire cose già dette da altri colleghi. Mi pare di partire dai beni oggetto di tutela da parte di questa norma che ci accingiamo ad approvare stasera; beni relativi ai diritti inalienabili, inviolabili, ai diritti della persona. Molti colleghi hanno messo in evidenza che si è intervenuti a legiferare su questa materia in presenza di un vistoso allarme sociale che si era creato qualche tempo fa su fatti specifici. Qualcuno lo ha detto con accezione negativa. Credo che il compito del Parlamento, del legislatore sia esattamente quello di dare risposte quando i problemi si pongono. Quindi, se in un determinato momento della nostra storia democratica, qualche mese fa, si è determinata una situazione di allarme sociale tale da richiedere necessario l'intervento del legislatore, credo che sia un buon legislatore quello che interviene non fuori tempo o magari tardi, ma quando è necessario che lo faccia. Si è pensato di usare lo strumento del decreto-legge. Sono qui a sostenere la giustezza di quella scelta, cioè dell'uso del decreto-legge, perché mi pare che nell'intervento del presidente Andreotti in discussione generale generale siano emersi gli elementi in base ai quali la necessità e l'urgenza giustificassero il ricorso al decreto-legge. Non faccio riferimento al «Taci! Il nemico ti ascolta», che ha citato il presidente Andreotti, ma all'indagine che lui ha svolto e che, secondo me, se la facessimo tutti quanti assieme, darebbero lo stesso risultato: quella sulla ancora assenza nel massimario di condanne per violazione del segreto istruttorio, nonostante vi sia una previsione normativa che risalga a diversi anni fa. Credo che il presidente Andreotti abbia ben incentrato la necessità necessità alla base della decretazione di urgenza in un momento in cui l'allarme sociale richiedeva un intervento che tranquillizzasse, che mettesse il cittadino in condizione di sentirsi tutelato attraverso i propri rappresentanti, cioè attraverso i legislatori. è stato poi un lavoro in Commissione - lo voglio dire con chiarezza - grazie all'abilità, alla bravura, alla comprensione del presidente Salvi, che ha portato al risultato che stiamo verificando qui stasera: quello cioè di avere la stragrande maggioranza del Senato d'accordo su un testo. Eppure, non era né facile è avvenuto nonostante - lo dico perché ieri c'è stata - qualche rapida incursione governativa che ha corso il rischio di far venire meno il clima che si era creato all'interno della Commissione che probabilmente poi avrebbe raggiunto, così come faremo tra poco quando voteremo il disegno di legge, gli obiettivi che il Governo intendeva raggiungere e che, per quanto riguarda noi senatori dell'Italia dei Valori, intendevamo raggiungere: tre senatori - lo dico per il senatore Castelli

volevamo raggiungere erano quelli di correggere - lo ha detto già prima di me in discussione generale il senatore Casson - qualche errore in cui il Governo era incorso in relazione a chi dispone; infatti, la previsione che il pubblico ministero possa disporre un qualcosa (lui parte nel procedimento), probabilmente era un errore che avrebbe viziato di incostituzionalità l'intero provvedimento. Era quindi opportuno con un giudice, nel caso di specie il giudice per le indagini preliminari, colui che ha il potere di disporre la distruzione. Abbiamo posto freno ad un errore che probabilmente, per la fretta con cui era stato steso questo provvedimento, non ci si era avveduti di commettere, così come pure al fatto che la stessa intercettazione, illegalmente raccolta, finisse con il diventare oggettivamente prova di un reato, quindi corpo del reato, per cui occorreva intervenire - così come con l'emendamento proposto dalla Commissione, che su quello che finiva con l'essere un vero e proprio corpo del reato rispetto al quale una qualche maggiore attenzione andava posta. Ad ogni modo, siamo riusciti a fare un buon lavoro, con un confronto sereno e leale in cui, anche quando non abbiamo accolto suggerimenti o osservazioni che venivano da altri colleghi, lo abbiamo fatto però riconoscendo agli stessi valenza tale da poter servire in un dibattito che io credo non finirà qui stasera su tali questioni. Mi sembra pertanto di poter dire - lo diceva nel suo intervento il senatore Caruso - che tutto è bene quel che finisce bene. Credo che voteremo un provvedimento che sicuramente per tempestività e per come è articolato raggiungerà gli obiettivi che ci siamo prefissati. Non mettiamo la parola fine su questa vicenda, ma abbiamo messo un puntello tale che ci consente probabilmente di essere una Nazione

Quando il 22 settembre scorso il Governo ha emanato il decreto-legge n. 259, recante disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche, sono state quasi all'unanimità riconosciute la necessità e l'urgenza di questo provvedimento. In particolare, il decreto è stato salutato positivamente da tutte le parti politiche e nessuna ne ha messo in discussione i requisiti costituzionali. Questo anche perché, come è noto, il Governo aveva, con correttezza e sensibilità istituzionale, tenuto conto della delicatezza della materia trattata, aveva preventivamente informato autorevoli esponenti dell'opposizione delle linee di intervento e delle misure contenute nel decreto stesso, come ha ricordato in Aula, ad inizio seduta, il relatore Salvi, presidente della Commissione giustizia. Questo non ha impedito una seria ed approfondita analisi del contenuto normativo del provvedimento, nel momento in cui se ne decideva la conversione in legge. Il lavoro svolto dal Senato, nel quadro della tutela della *privacy*, si è indirizzato prevalentemente nel garantire un migliore bilanciamento degli interessi costituzionali in gioco, nel condividere l'obiettivo del rafforzamento del contrasto alla detenzione di materiali abusivi e di *dossier*, la cui formazione va impedita anche con un serio inasprimento delle pene, tra l'altro previsto dal decreto per chi dovesse rendere pubblici i contenuti del lavoro di dossieraggio illegale. Ci si è concentrati nella definizione o nella migliore specificamente di elementi che potessero garantire anzitutto la parte offesa, anche in termini di risarcimento. Se le operazioni di distruzione avvengono con modalità tali da assicurare il rispetto di tutte le garanzie necessarie al pieno esercizio dei diritti di difesa, preferibilmente nel contraddittorio delle parti, davanti al giudice e, comunque, con garanzie di riservatezza, si può allora affermare che il lavoro di affinamento del testo ha raggiunto un obiettivo, direi, assai importante. Sul punto si è avuta ampia convergenza, essendo obiettivo comune quello di prevedere particolarità di conservazione del materiale per lo stretto tempo di attesa della realizzazione del contraddittorio sulla sua distruzione. La finalità del decreto-legge era quindi non solo e non tanto quella di fornire una prima risposta ad una emergenza sul fronte di garanzia della*privacy*, ma anche di offrire garanzie per tutti - com'è stato contrassegnato in Aula da diversi colleghi, tra cui il senatore Tibaldi e la senatrice Boccia compresa la collettività, nella trattazione dei dati protetti da parte di chiunque. È, quindi, un provvedimento di tutela generale quello che siamo chiamati a convertire in legge. Certamente, nell'effettuare una valutazione sul testo, non si può prescindere dalle condizioni - queste, sì, davvero straordinarie e preoccupanti - che ne hanno determinato l'emanazione. A partire da una lunga e complessa indagine della magistratura e grazie ad un coraggioso lavoro giornalistico d'inchiesta, è emersa una realtà illegale consolidatasi nel corso di almeno un decennio e talmente ramificata da far asserire a qualcuno che la stessa democrazia era a rischio. La democrazia ha, per fortuna, strumenti d'intervento ancora efficaci: una magistratura indipendente ed autonoma, una libera stampa ed anche un Parlamento, che è chiamato a varare tutte le misure idonee ad evitare che il sistema illegale scoperto abbia a perpetuarsi o a ripetersi. Non dobbiamo mai dimenticare che ciò con cui ci si deve misurare è un fatto di portata difficilmente comparabile con analoghe vicende nella storia repubblicana, se non altro per ampiezza e caratteristiche del sistema illegale e delle sue «vittime». Se, infatti, per un decennio sono stati abusivamente raccolti dati riguardanti migliaia di cittadini, appartenenti alle più svariate categorie (dall'operaio al *vip* della finanza, dal politico alla *soubrette* dello spettacolo, dal calciatore al dipendente aziendale o al semplice cittadino «cliente»), vuol dire che si va ben oltre un ristretto gruppo di soggetti, in una specie di organizzazione affaristica piramidale, annidatasi all'interno di una grande impresa di telecomunicazioni, per altro dichiaratasi parte lesa. I giudici che hanno vagliato, nell'ambito delle indagini preliminari, le evidenze raccolte dal pubblico ministero hanno infatti parlato di un vero e proprio sistema, che, grazie ad una consistente, per non dire enorme, disponibilità di denaro, commissionava e gestiva un complesso di indagini parallele. Il pagamento di attività corruttive e l'utilizzo di opache collaborazioni, finanziate con fondi drenati alle imprese, sarebbero stati utilizzati per migliaia di intercettazioni telefoniche illegali (intendendo con tale termine la raccolta dei dati e dei tabulati), pedinamenti, sistemi di videosorveglianza e *software*, sfociati - quantomeno dal 1997 ad oggi - in un immenso archivio segreto, in cui si schedavano dipendenti, finanzieri, *manager* e politici. Ma oggi siamo chiamati a dirimere una questione che va ben oltre tale specifica vicenda, che è in fase di accertamento. Le parole di allarme democratico del presidente Prodi, allora, sono pienamente giustificate e devono far riflettere, ma questo ben al di là del singolo caso giudiziario, per quanto grave e preoccupante. Se è vero che per qualcuno è stato impossibile controllare al terminale SDI delle forze dell'ordine i precedenti di polizia del personale che sarebbe stato assunto e che venivano compiuti e reiterati accessi abusivi al sistema dell'anagrafe tributaria (nell'ambito di una pluralità di operazioni dai nomi fantasiosi, che consistevano nell'illegale incursione all'interno delle migliori banche dati informatiche, con tanto di tariffario per la compravendita dei dati e dei tabulati telefonici di ignari cittadini: da 250 fino ad un massimo di 1.500-2.000 euro), com'è possibile non intervenire con norme adeguate? Se è vero che i dati sensibili (numeri di telefono, riferimenti bancari e vite private dei singoli cittadini) venivano raccolti in *dossier* dai nomi in codice e con sistemi di schedatura e controlli sul territorio attuati da una pluralità di soggetti (investigatori, pubblici dipendenti pubblici dipendenti infedeli, eccetera) che per denaro vendevano informazioni, è evidente che vi è una grave falla nei sistemi di controllo, anche se in recenti audizioni così è stato, ma sono ancora in corso in Commissione giustizia - molti esperti e vertici aziendali hanno offerto rassicurazioni (tutte da verificare). Che si trattasse di un dossieraggio illegale lo prova il fatto che tale documentazione non doveva in alcun modo essere conservata, tanta che «a partire da un certo momento ha cominciato addirittura ad essere bruciata», come si legge nell'ordinanza del GIP. Ma se un caso specifico ha suscitato allarme nell'opinione pubblica, dovere del Parlamento è di approvare leggi generali capaci di prevenire simili situazioni nel futuro e di regolare in modo efficace la materia. si è, dunque, posto come primo obiettivo quello di sradicare la decennale prassi di schedare, spiare, catalogare i cittadini di volta in volta ritenuti di interesse e i loro numeri telefonici. Il decreto modifica il codice di procedura penale per colpire questo tipo di attività illegali, introduce nuovi reati e regola alcuni rapporti civilistici in tema di risarcimento del danno. Per questo, con una modifica apportata dalla Commissione e votata all'unanimità (a parte alcuni voti contrari) all'interno di questo Parlamento, siamo in qualche modo

nel corso dell'esame parlamentare si è convenuto, ad esempio, che la distruzione di questo materiale, che non sarebbe mai dovuto esistere, rappresenti il punto centrale dello stesso provvedimento poiché l'illegalità della formazione, anche per garantire il diritto della difesa, può essere stabilita nel contraddittorio delle parti. Si è pensato fosse più utile individuare un meccanismo per cui fosse il giudice dell'udienza preliminare, con decreto motivato, a disporre la distruzione. È, dunque, ragionevole pensare ad un sistema che assicuri l'immediata secretazione del materiale e il divieto di utilizzo dello stesso, il che non inibisce immediatamente e del tutto un utilizzo a fini investigativi del corpo del reato. Mi resta però un'ultima cosa da dire in chiusura. Fermo restando il nostro voto favorevole, rimane un problema. Si è parlato e discusso di intercettazioni illegittime, ma quante volte le intercettazioni cosiddette legittime diventano illegittime nell'uso che ne viene fatto da tutti i soggetti che abbiamo citato ampiamente all'interno di questo Parlamento? Credo che questa sia la riflessione che tutti ci dobbiamo porre

Signor Presidente, il gruppo UDC ha preferito non svolgere alcun intervento nell'ambito della discussione generale e di riservare parte del tempo (ovviamente, non intendo parlare per tutto il tempo di cui l'UDC dispone) per cercare di dire che cosa, a nostro giudizio, riteniamo sia avvenuto e quale insegnamento politico per il futuro riteniamo di cogliere. Questa è una vicenda di grande rilievo. Occorre comprendere che è stato predisposto un decreto-legge con il consenso di tutti i *leader* dei Gruppi di opposizione. Il fatto politico di grande rilievo è avvenuto nel momento in cui è stato adottato il decreto-legge

e non è la prima volta. Ma lo ha potuto fare perché era esploso un caso straordinario, una rivoluzione nell'opinione pubblica generalizzata, prevalentemente parlamentare ma non soltanto, in seguito alle cosiddette notizie delle migliaia di intercettazioni Telecom. La saldatura di questi due fatti ha consentito l'adozione del decreto-legge. Che cosa si è ottenuto attraverso quel decreto-legge, altrimenti non capiamo di cosa stiamo discutendo noi oggi, a mio giudizio? è ottenuta l'immediata scomparsa dai giornali della Repubblica della vicenda delle intercettazioni illegittime. Si è ottenuto un fatto politico, non un fatto giuridico.

Successivamente, è cominciata una vicenda giurisdizionale, procedurale, politica e parlamentare molto complicata. Il decreto‑legge è stato presentato al Senato aveva la copertura politica dell'accordo generale. Occorreva verificare se vi erano le condizioni processual-parlamentari per un'intesa generale. Pertanto, l'oscillazione che ha avuto ieri il Governo,

perché stava mettendo in crisi la premessa politica del decreto-legge, cioè la ricerca dell'intesa. Se gli emendamenti che il Governo ha presentato avessero avuto la possibilità di realizzare un'intesa larghissima, nessuno avrebbe avuto nulla da obiettare. Però in quel momento

della vicenda delle intercettazioni illegittime, quanto per il fatto che quel decreto-legge aveva prodotto un risultato straordinario mediatico, quello della cancellazione della vicenda dai giornali,

ma dal punto di vista giuridico e parlamentare è il testo della Commissione: è la saldatura tra l'intesa politica che regge il decreto-legge e l'intesa tecnico-costituzionale che ha retto la Commissione. Si realizza così un accordo che altrimenti non sarebbe stato

perché abbiamo alle spalle un passaggio di grande rilievo, al quale sono rammaricato che la stampa italiana non abbia dato il significato che meritava, quello che ha consentito di tenere in vita, non più sospesi, due

e l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione disciplinare. Questi due pilastri intatti hanno rappresentato un piccolissimo ma significativo avanzamento verso una posizione che ha consentito

fine della cosiddetta Prima Repubblica), dalla linea dello scontro totale con l'ordinamento giudiziario (nel quale sostanzialmente il Parlamento perde il potere legislativo, perché nello scontro

formula di estremo significato costituzionale) e di Regioni (per le quali altrettanto si predica l'autonomia in Costituzione) si cerchino in questa legislatura intese tali da far comprendere che chiunque vince le elezioni non ha la totalità del potere legislativo, né in materia religiosa, né in materia giurisdizionale, né in materia istituzionale regionale. Questo è il messaggio importante che dal Senato sta venendo fuori. Tale messaggio richiede che il Governo della Repubblica sposi la linea dell'intesa istituzionale, non come inciucio, ma come questione istituzionale di fondo, laddove necessaria. Questo è il merito che riconosco al mio antico amico

dico «in particolare» per la tutela che il sistema proporzionale giustamente prevede per i singoli Gruppi - la volontà di cercare l'intesa su queste tre questioni di fondo, senza alterare la cultura bipolare che è al fondo della nostra azione politica

in questi giorni in materia di giustizia al Senato. Cercherò di spiegare perché. Mi sembra che riusciamo a ottenere degli accordi quando non ci sono sul tappeto i problemi reali o comunque i problemi più importanti. È accaduto sulla questione dell'ordinamento giudiziario, dove la maggioranza ci ha concesso - o è stata obbligata dalla forza dei numeri - di discutere e di arrivare ad un compromesso su due decreti legislativi significativi, ma poi ha fatto muro e quadrato sul decreto legislativo fondamentale, o almeno quello che l'ANM ritiene fondamentale perché contiene due *totem* negativi per l'Associazione stessa, cioè la cosiddetta separazione delle carriere e la progressione in carriera basata sulla meritocrazia, termine che i magistrati - quanto meno la loro rappresentanza - evidentemente aborriscono. Mi pare che anche oggi si sia in qualche modo ripetuto questo copione, perché c'è un esimio esponente politico di questa parte della storia politica del Paese, Silvio Berlusconi, che spesso si rifà al teatrino della politica. Bene, colleghi, io sono convinto che noi oggi siamo stati tutti attori di questo teatro, tra queste quinte, perché, come ripeto, e ne sono sempre più convinto stante l'andamento del dibattito, noi abbiamo legiferato sul nulla. sul nulla. Infatti, non esiste un solo atto concreto - vorrei che qualcuno me lo esternasse e me lo mostrasse - che dichiari che in passato o nel presente vi siano state delle intercettazioni acquisite illecitamente e illegalmente. Non vi è neanche un atto concreto, quindi noi ci siamo preoccupati di una questione meramente virtuale. Poi c'è qualcuno, come il senatore Formisano, che per tutto ciò si è sentito più europeo: beato lui, io francamente non riesco a capirne la ragione. È evidente: abbiamo fatto del teatro, abbiamo fatto finta di legiferare su un tema cruciale come quello della propalazione delle intercettazioni parlando d'altro e non abbiamo assolutamente affrontato il tema reale. D'altro canto, basta vedere anche i mezzi. Quando il Governo vuol parlare di qualcosa che non c'è, di un mondo virtuale, allora affronta il tema con un decreto-legge e quindi fa un'operazione mediatica che, a mio parere, va smascherata, perché poi, in politica, quello che conta non è ciò che è vero ma ciò che sembra vero e ciò che percepisce l'opinione pubblica. Colleghi, l'opinione pubblica ha percepito che il Governo, con grande rapidità, velocità ed efficacia, al contrario di quanto abbiamo fatto noi nella scorsa legislatura, ha affrontato lo scottante tema delle intercettazioni e della loro propalazione sui giornali, e quindi l'immagine data al Paese è stata: il Governo Berlusconi non è stato in grado di far nulla; guardate invece il governo Prodi

Come si fa ad affermare che bisogna immediatamente distruggere un corpo di reato? È una bestialità che capisce chiunque, ma forse non chi ha scritto il decreto. L'abbiamo messo a posto dal punto di vista formale, perché non potevamo fare altro; forse sarebbe stato più dignitoso lasciarlo decadere perché è ovvio che non vi è alcuna urgenza su questo tema, dato che non esiste nulla su cui intervenire. A questo però, ribadisco il mio dubbio che resta nella mente di molti, compresi alcuni esponenti della maggioranza, sulla motivazione per la quale si è agito così rapidamente un certo giorno su questo tema. Forse è stata fatta un'altra seduta spiritica in cui, anziché quella su via Gradoli, è arrivata al Governo Prodi qualche altra informazione dal bicchiere. c'è stato un momento in cui occorreva bruciare tutto, bisognava mandare tutto al rogo rapidamente, altrimenti chissà che cosa sarebbe successo. Il presidente Prodi ha parlato addirittura di contagio, c'era un contagio. E allora, alla stessa stregua dei monatti manzoniani, bisognava bruciare tutto affinché la peste non dilagasse. Peccato che nessuno riesca a dimostrare dove sia questa peste,

ci sono delle testimonianze, rese in Commissione dagli esponenti della Telecom, che potrebbero anche mentire ma, fino a prova contraria, in Commissione si dice la verità, che ci dicono che è impossibile tecnicamente acquisire illecitamente queste intercettazioni senza lasciare una traccia telematica.

mobile qual piuma al vento a seconda delle maggioranze e dei Presidenti. Come mai secondo la Costituzione, che è sempre la

la storia di questo decreto è già stata narrata a più voci. Quindi, non mi dilungherò, data anche l'ora.

specialmente in campo Telecom. Il decreto inviava un messaggio netto e rapido al Paese sul contrasto all'illegalità di queste forme d'indagine.

essi non potranno essere poi contrastati con molta *nonchalance* né dall'Associazione nazionale magistrati, né da altri settori. Infatti, essi rivelano un accordo parlamentare quasi unanime. questo decreto legifera sul nulla, come ho già detto. C'era l'emergenza dei fascicoli della Telecom, ma c'è sempre la possibilità che ci siano anche delle telefonate intercettate illegalmente e non c'è dubbio che il legislatore deve anche essere preveggente, deve anche legiferare per il futuro. Ritengo, quindi, che abbiamo anche predisposto uno strumento valido

Se avessimo assecondato queste pulsioni, avremmo determinato un passo avanti verso l'imbarbarimento della vita civile, politica ed economica di questo Paese. Invece, abbiamo stabilito che dalle intercettazioni e dalle fascicolazioni illegali non si può trarre niente di utile, se non la prova per perseguire chi ha effettuato queste intercettazioni - nel rispetto del contraddittorio delle parti e del giusto processo disposto da un giudice

per quei reati specifici, cioè della intercettazione e fascicolazione illegale, a carico ovviamente di chi le ha fatte e con la salvaguardia delle persone offese che, appunto, hanno un ruolo anche anche nella fase procedimentale della distruzione. Credo che anche il problema della responsabilità civile sia stato risolto in modo abbastanza brillante e ne va dato atto al collega Caruso, che ha trovato la formula perché un decreto di distruzione potesse essere portato davanti al giudice civile. questo senso abbiamo fatto un passo molto importante. Per quanto riguarda poi il bilanciamento tra il dovere dello Stato di tutelare la *privacy*, la riservatezza dei cittadini, e il dovere della stampa di tutelare la libertà di stampa, credo che si sia raggiunto un buon equilibrio.

per cui il destinatario, leggendo il giornale, può prendere il treno o l'aereo ed andarsene via. Ritengo che questa notizia non bilanci

base delle dichiarazioni di Buscetta, alla fine dell'istruttoria del maxiprocesso, perché la notizia era stata raccolta da un settimanale che sarebbe uscito di lì a poco, dando, appunto, ai mafiosi l'annunzio che era meglio porsi porsi in salvo, invece di aspettare a casa i Carabinieri. Quindi, fummo costretti in una notte a scrivere e firmare tali ordini di cattura e quei mafiosi furono catturati. Non credo ci fosse una necessità, un'opportunità, un diritto dei cittadini di sapere che quei mafiosi

Signor Presidente, colleghi, Alleanza Nazionale voterà a favore del provvedimento, certamente con quell'approccio laico, problematico ma costruttivo con il quale ha seguito i lavori della Commissione ed ha contribuito a rendere dignitoso il testo, decorosa una legge e fattibile un'ipotesi presentata con superficialità dal Governo.

Aggiungo considerazioni riassuntive e finali, principiando da una di carattere generale, che mi vede dissenziente dall'intervento dell'ex ministro Castelli: la giustizia è una necessità della società, non è un'opzione personale o soggettiva e quando sul terreno della giustizia si incontrano culture e soggetti diversi, il cammino che si riesce a percorrere è sempre un cammino virtuoso. Sul terreno della giustizia, nel corso di questa legislatura, abbiamo conseguito finora due risultati che ritengo positivi

ma anche e soprattutto per quella capacità di ascolto e di addizione che noi della Casa delle libertà abbiamo saputo portare in ogni momento del percorso. Mi rendo conto che quando abbiamo esaminato con attenzione i decreti legislativi dei quali si voleva posporre l'entrata in vigore all'anno e quando ci siamo approcciati a discuterne in termini realistici, siamo stati noi dell'opposizione, certamente insieme alle intelligenze recettizie che vi sono anche dall'altra parte dello schieramento, a determinare i punti della convergenza.

della Costituzione. Il nostro intervento ha determinato finalmente nell'ordinamento giudiziario varchi e aperture che non erano concepibili soltanto qualche mese fa.

È un parere aperto. È un parere colloquiale. È un parere, come è previsto dalla legge, quando il Ministro ne fa richiesta, come in questa occasione. Non si tratta di proclami da quarta Camera che il Consiglio superiore della magistratura, anche nel periodo in cui ne facevo parte, lanciava nei confronti delle forze politiche e del Parlamento, sì da determinare spesso condizioni di subordinazione psicologica. psicologica. Quando sul tema della giustizia riusciamo a far sì che il Governo retroceda dal suo proposito di posporre l'entrata in vigore dei decreti relativi per oltre un anno e costringiamo le forze della maggioranza e del Governo, si può capovolgere l'ottica con cui l'ottimo senatore Castelli vede le cose. È vero che vi è un teatrino della politica, ma - certamente il senatore Castelli non lo ignora - un grande giurista del Settecento, che ha scritto il «*Theatrum veritatis et iustitiae*», ha spiegato come si svolge e come nasce il processo, il teatro delle verità, su cui abbiamo costruito questo percorso, portando la maggioranza a consentire che finalmente i magistrati potessero sentirsi uguali a tutti noi con l'entrata in vigore della legge sugli illeciti disciplinari. Avete letto i comunicati pervenuti dall'Associazione nazionale magistrati? Avete sentito dei tavoli che si sono aperti, sia pure per vili questioni pecuniarie, a Palazzo Chigi, come puntualmente avviene? Qual è stato il risultato? Vi è stata la resa, come spesso è avvenuto? Vi è stata la fuga, come spesso è avvenuto? O vi è stato piuttosto un atteggiamento di responsabilità doverosa da parte di tutti noi? Per la prima volta, in queste due occasioni, i soggetti si sono guardati attorno rispettandosi con dignità, ognuno al suo posto. Certo, avevamo e abbiamo il dovere di sentire la voce della magistratura. Avevamo e abbiamo il dovere di rispettare la magistratura come corpo autonomo, indipendente, imparziale e, secondo l'articolo 111 della Costituzione, oggi anche terzo; vi è, infatti, una differenza non lessicale tra imparzialità e terzietà. Ma una cosa è ascoltare questa voce e un'altra è, invece, discutere in condizioni di minorità. Abbiamo discusso in condizioni di grande parità e per la prima volta ci siamo sentiti, nel corso di questi anni, finalmente in grado di portare un contributo notevole nel corso del dibattito. Questo è un aspetto positivo che non deve essere trascurato. Certo, in questa occasione si è verificato un fatto assai grave. Colleghi, ho ascoltato con molta attenzione le parole sagge del presidente Andreotti, del presidente Andreotti, il quale ha fatto riferimento ad una necessità psicologica nella risposta che il Parlamento offre con l'approvazione di questa legge. Ricordiamo qual è la genesi di questa legge. Essa è nata su basi politiche ed emotive.

Lasciamo stare se si trovano le intercettazioni abusive: si sono trovati i tabulati abusivi. Lasciamo stare se la virtualità si determinerà domani in concretezza. Abbiamo comunque avuto tutti la sensazione che le notizie potessero corrispondere al vero e che a quelle parole potessero corrispondere i fatti. i fatti. Tutti siamo convinti che possano determinarsi quelle certezze, quei fatti, quei comportamenti e quelle condotte trasgressive. È stato un momento difficile: non si trattava della patologia che segue al processo penale, perché quella è patologia.

non si trattava di una patologia nella fisiologia del processo penale. Si trattava piuttosto di una gravissima forma di patologia che abbiamo vissuto sotto i nostri occhi: non c'erano giudici, cancellieri, avvocati, mediatori degli uffici giudiziari. No. C'erano, dall'altra parte, gruppi di potere, probabilmente consorterie criminali, che si organizzavano per captare conversazioni, per intervenire in maniera interferente nella vita dei cittadini, per coglierne gli aspetti più remoti, ai fini certo di un'utilizzazione illecita futura, perché ciò non si fa per gioco o per *voyeurismo* politico, ma per altri e chiari motivi. Di fronte a questa situazione gravissima, a questa patologia che ha ammorbato il nostro Paese e di fronte soprattutto, signor Presidente e onorevoli colleghi, ad una confusione di ruoli nella società e ad una costante abdicazione dei valori, era necessario dare una risposta.

qualche volta di sciatteria metagiuridica con cui è stato scritto, poco importa. Importa che ci sia stato fornito lo strumento attraverso cui anche noi abbiamo contribuito, in maniera decisiva e determinante, a far sì che perlomeno si sappia che, di fronte a questa massiccia patologia, c'è

Se abbiamo fotografato delle trasgressioni, abbiamo nello stesso tempo posto una grande deterrenza pedagogica per il futuro. Ecco perché questo intervento risponde alle necessità dall' emozione del momento ma si pone, come giustamente diceva il presidente Andreotti, nel quadro di una necessità psicologica a cui - nella società e per la società - il Parlamento ha risposto. E abbiamo risposto bene,

Aula. Si è insistito moltissimo, a seguito delle sollecitazioni del collega Nitto Palma, su una modifica della procedimentalizzazione all'articolo 3. Si tratta di un intervento calligrafico celestiale,

garanzie, della celerità e dell' aspetto risarcitorio, hanno determinato certezze. Noi senatori della Casa delle libertà e di Alleanza Nazionale crediamo di aver dato in queste ore e in questi giorni una dimostrazione di obiettività, di stile e di responsabilità.

per alcune ragioni, che riassumerò rapidamente perché non voglio far perdere tempo all'Aula. L'ex ministro Castelli ha posto alcune domande a cui sarebbe opportuno dare risposta, non ha posto tutte le domande alle quali occorre rispondere. Se c'è una questione che ho condiviso tra quelle trattate nell' intervento del senatore Buccico, è quella riferita all'emozione che ha dettato la necessità di varare questo provvedimento. Mi chiedo però se questa emozione abbia trovato risposta, se oggi i cittadini siano rassicurati. Vorrei poterlo dire con la stessa certezza dei miei colleghi. un provvedimento varato troppo in fretta, diceva il senatore Salvi, troppo *bipartisan*, senza probabilmente dare alcuna risposta. anche se mi rendo conto di dire una cosa che ha una sua gravità, quali siano stati gli interlocutori a conoscenza delle intercettazioni disposte dal gruppo criminale che operava all'interno di Telecom; non so ancora se il dottor Tronchetti Provera ne fosse a conoscenza; non so quali fossero gli interlocutori politici, in quanti, in quali partiti e a quali livelli ve ne fossero del dottor Tronchetti Provera; quanti fossero a conoscenza di intercettazioni e, quindi, se non sia stato per questo che si sia deciso di distruggere tutto, perché chi legge le intercettazioni, teme ve ne siano in circolazione su di sé ed ha interesse a distruggerle tutte. Ecco perché, Presidente, ho qualche preoccupazione che, in realtà, non venga mai alla luce lo scandalo dello spionaggio politico nelle sue responsabilità. Mi è dispiaciuto il voto dell'Aula, anche se voglio apprezzare il voto favorevole del presidente Salvi all'emendamento presentato. Apprezzo il voto favorevole dei Gruppi che hanno contribuito, comunque, alla discussione. Credo che dobbiamo fare ancora dei passi in avanti. Manca dell'altro, potrei dire, a questo decreto. Lo ritrovo negli emendamenti bocciati del senatore Castelli. Credo che

Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, Forza Italia voterà favore del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 259. C'è uno sport molto diffuso in Italia: la pubblicazione di intercettazioni legittime, utile alla lotta politica, a sporcare l'immagine di tanti soggetti, ad innescare una serie di processi mediatici, in piazza in cui si emette già comunque una condanna o si danno patenti infami a persone che, comunque, non potranno mai essere ripagate, neppure dalla sentenza più ampiamente assolutoria. È uno sport diffuso, cui si aggiunge un'ulteriore patologia: quella di una ipotesi, di una possibilità di intercettazioni illegittime, fatte assolutamente al di fuori di ogni o qualsiasi forma di autorizzazione e controllo da parte del magistrato, semplici oggi perché il progresso tecnologico consente facilmente di accedere alla possibilità di intercettare utenze fisse, ma anche utenze mobili. Si sono verificate? Ci sono state? È vero, come qualcuno sostiene, che è stata tutta una invenzione dei *media* e dei giornali? Certamente si è innescato uno psicodramma, cui ha partecipato anche il Presidente del Consiglio, il quale ha dichiarato di essere stato anche lui spiato. Finalmente forse, si è potuto attribuire la patente di vittima, mentre invece è solo il responsabile di tutti i danni ed i disastri che stanno avvenendo in questo Paese a causa della conduzione del suo Governo! Tuttavia, si è innescata una vicenda che ha reso necessaria l'emanazione di un decreto-legge, indispensabile ad evitare i rischi di questa propalazione assolutamente illegittima; i rischi che questi atti, sequestrati nell'ambito di un processo penale, potessero comunque essere depositati, divenire pubblici e, quindi,

di prevedere anche sanzioni per la detenzione di questo materiale, di arrivare ad una distruzione immediata e non ad una distruzione che avviene successivamente, che consente il deposito degli atti e, quindi, la pubblicità di essi e che ne consente la propalazione con tutto ciò che ne consegue. A questo punto, però, si innesca una danza strana, perché improvvisamente alle ore di ieri il Governo presenta un maxiemendamento che capovolge assolutamente l'impostazione data al decreto legge. Si parlava di autorità giudiziaria in modo indistinto, ma evidentemente ci si riferiva al pubblico ministero, si inserisce il GIP - poco male - ma soprattutto non si parla più di distruzione immediata; si parla di distruzione che avviene dopo il passaggio in giudicato della sentenza, cioè dopo svariati anni, ovvero dopo un anno dal deposito del decreto di pubblicazione, il tempo, cioè, necessario a che il contenuto dell'intercettazione se ne possa tranquillamente andare in giro e possa essere propalato senza difficoltà. Cos'è successo? Improvvisamente, dopo due ore, contrordine compagni! Il maxiemendamento viene ritirato. Allora la Commissione ha lavorato, e penso anche, tutto sommato, con un prodotto qualitativamente elevato, ad una soluzione mediana che inserisce nel sistema, da un lato una immediatezza nella distruzione ma dall'altro anche una serie di garanzie, indispensabili a far sì che le parti partecipino al procedimento di distruzione e che, evidentemente, possano verificarne l'avvenuto compimento. Le indagini possono essere comunque sviluppate anche per verificare chi ha realizzato le intercettazioni illegittime, perché in ogni caso ne rimane traccia attraverso i verbali di sequestro e attraverso il verbale di distruzione. Il contenuto di questi atti era assolutamente inutile ai fini delle indagini che comunque possono assolutamente proseguire. Qual è il panorama però che si trae da tutta questa vicenda? Il panorama è desolante; è il panorama desolante di un Governo privo di un indirizzo certo e che non ha chiarezza sull'indirizzo politico nel sistema giustizia, se cambia idea da un momento all'altro, con estrema facilità, tornando poi sul suo primo intendimento. Ci si può chiedere cosa sia successo, se ci siano stati eterocondizionamenti, se qualcuno è intervenuto. Il collega Di Lello ha detto che non si appassiona a questa vicenda e fa bene perché è una vicenda triste, e però lui stesso ha dato la chiave di lettura: sono state vinte le pulsioni giustizialiste di cui avrebbe voluto conservare questi atti per poter ripartire e ha dato quindi l'origine di questo immediato cambiamento di rotta del Governo, a cui è poi poi seguito l'ulteriore passo indietro. Il panorama è desolante perché c'è un Governo che non è neppure raccordato con la sua maggioranza che neanche sapeva della presentazione di questo emendamento. Il panorama è desolante perché poi, alla fine, questa maggioranza è una maggioranza tributaria della minoranza per le idee che hanno connotato non solo il precedente disegno di legge di sospensione quasi - non del tutto - della riforma dell'ordinamento giudiziario, ma anche di questo disegno di legge, se solo pensiamo che l'articolo 4 viene riscritto totalmente dal collega Caruso e che gli articoli 1 e 2 passano attraverso le indicazioni provenienti dai Gruppi della Casa delle Libertà. È un'ulteriore dimostrazione dell'assenza di idee a cui noi dovremo far fronte. Siamo una minoranza responsabile e pensiamo che il pianeta giustizia debba trovare soluzioni rapide e sarà nostra cura, nell'assenza totale di un indirizzo da parte del Governo, e anche di indicazioni

sono state sostanzialmente accettate per la riforma dell'ordinamento giudiziario, per quanto riguarda i due decreti delegati della procura e per la vicenda della materia disciplinare saranno sostanzialmente accettate anche per la separazione delle funzioni, considerate le dichiarazioni del Ministro e di eminenti colleghi della maggioranza. Allora, forti di questa certezza, di poter proporre delle idee valide, andremo avanti e saremo noi propulsione per la riforma della giustizia, a differenza di un Governo latitante e di una maggioranza assolutamente priva di idee.

quello che ci accingiamo ad approvare è un atto normativo necessario, un'iniziativa urgente, un primo passo per l'opera di bonifica di bonifica degli apparati e di moralizzazione della quale il Paese ha bisogno. Da quale vicenda nasce il decreto-legge che stiamo discutendo? Vi è stata, nei mesi scorsi, un'indagine giudiziaria delicata, che ha dato luogo all'emissione di una serie di provvedimenti di custodia cautelare: nella complessa e vasta ordinanza di cui la stampa ha dato notizia vi era la ricostruzione di gravi attività illecite. Alcune questioni, aperte di fronte a noi e all'attenzione del Paese, nascono da quell'indagine e si possono mettere a fuoco se si legge quell'ordinanza. A dirla in breve, si era costituito, nella più grande azienda del Paese, un centro di potere occulto, dedito alla raccolta di informazioni, documenti e dati sensibili alla redazione di *dossier*, contenenti informazioni e pseudo-informazioni*,* i quali potevano servire per attività calunniose, per la diffamazione di terzi oppure per contenere informazioni su persone, acquisite illecitamente ed il cui uso, proprio in ragione di tale acquisizione, non poteva che essere illecito. Questo gruppo, che operava nell'ambito di una grande azienda, o dipendeva dal vertice Telecom o ha truffato l'azienda. Ci domandiamo: a chi obbediva? Quali erano i fini che perseguiva? Sul punto, signor Presidente, le questioni sono tuttora aperte ed è necessaria una risposta: attendiamo un accertamento delle responsabilità da parte delle autorità giudiziarie competenti. Ma vi è, di fronte ad una situazione così complessa e piena di negatività, un compito, un dovere che spetta ed incombe sulla politica e che non può esaurirsi, a nostro giudizio, nel decreto‑legge, pur importante, che stiamo in queste ore discutendo. Vi era, alla base di tali attività illecite, una sinergia tra funzionari dell'azienda telefonica, investigatori privati e pubblici ufficiali infedeli: ed è di questa terza categoria che abbiamo il dovere di occuparci con particolare attenzione e impegno, perché vi sono dati sensibili ed informazioni che non possono essere acquisiti senza la collaborazione e l'intervento di pubblici ufficiali infedeli. Questo è un nodo da sciogliere, è un problema da risolvere. Ad essere bersagliati dall'attività spionistica e dalla creazione di *dossier* che si realizzavano attraverso tale tipo di collaborazione, sono stati esponenti del mondo imprenditoriale e della politica, con un effetto duplice: inquinare la competizione economica (questa era la funzione dei documenti illecitamente raccolti) ed il sistema politico.

perché l'inquinamento della competizione economica e del sistema politico riguarda le condizioni di vita della nostra società e della nostra democrazia. Noi dobbiamo sbarrare la strada all'inquinamento, alle attività illecite, allo spionaggio, alla manipolazione dell'economia e della politica perché è nell'interesse della collettività e dei cittadini. Vi erano, tra l'altro, informazioni e dati sensibili che si riferivano a lavoratori dipendenti, oppure a giovani che avevano presentato domanda di assunzione alla Telecom. Poiché anche in questo caso questo caso ci troviamo di fronte ad una gravissima violazione di legge, anche per loro deve valere la regola della distruzione. Non c'è alcuna giustificazione per la schedatura dei lavoratori e non c'è rischio di terrorismo, non vi sono motivi fantomatici che possano giustificarla nei termini in cui noi l'abbiamo conosciuta attraverso le notizie e le informazioni date dalla stampa in queste settimane. Il decreto-legge stabilisce che questi documenti, questi dati sensibili, queste informazioni, insomma che l'insieme di tutta quella spazzatura che era stata raccolta e che doveva essere messa in circolazione, venga distrutta secondo regole tali da garantire che non vi sia alcun colpo di spugna sulle responsabilità di coloro che hanno acquisito quei documenti, che hanno messo insieme quelle informazioni, che hanno utilizzato quei dati sensibili a fini di inquinamento dell'economia e della politica. Dobbiamo sapere chi sono, certo. Ma intanto cominciamo a creare le condizioni perché la spazzatura non sia messa in circolazione sia messa in circolazione e affinché i responsabili possano essere perseguiti. Noi, proprio a proposito del tema della distruzione dei documenti e delle informazioni, abbiamo spiegato al Governo che gli emendamenti presentati ieri non erano accettabili in quanto differivano in modo irragionevole con quella distruzione necessaria che, del resto, era l'obiettivo che si era voluto perseguire attraverso lo strumento del decreto-legge rispondente ai requisiti di necessità ed urgenza. Il Governo, proprio sulla basa delle nostre critiche, delle critiche venute dalla maggioranza, ha compiuto la scelta corretta di ritirare quegli emendamenti e di rimettersi al Parlamento. Noi abbiamo stabilito che vi sia distruzione nel più breve tempo possibile con garanzie per le parti interessate e, in particolare, per chi è stato vittima delle attività spionistiche dei *dossier* calunniosi; abbiamo stabilito che sia un giudice terzo a decidere e a disporre la distruzione; che il contenuto di questi documenti non possa essere in alcun modo utilizzato; che chiunque, consapevolmente, li detenga sia punito con una pena da sei mesi a quattro anni e abbiamo anche stabilito che, nel caso di pubblicazione, coloro ai quali gli atti o i documenti fanno riferimento hanno diritto a chiedere una riparazione pecuniaria. Vorrei dire, dopo le parole in certi tratti inutilmente polemiche del collega Centaro, che l'Ulivo è stato protagonista del raggiungimento di questa intesa e aggiungo, proprio perché non mi piacciono le polemiche senza senza senso e fuori luogo, che nessuno di noi, né noi né i colleghi del centro-destra che hanno partecipato al lavoro in Commissione, ha rinunciato alle proprio valutazioni di partenza, al proprio punto di vista. Non c'è bisogno, collega Centaro, per rivolgersi alla propria opinione pubblica di fare qui in Aula la faccia feroce e di attaccare il Governo e la maggioranza. Stiamo concludendo un lavoro che abbiamo condotto insieme. Ci sono tanti argomenti su cui questo non è uno di essi. O forse, ho capito male e quindi il voto che vi accingete a dare non è un voto convinto. Ma non lo credo, perché ho visto che in Commissione la convergenza si realizzava e che abbiamo potuto lavorare utilmente. Siate tranquilli, il bipolarismo è salvo, il contrasto tra noi e voi rimane tutto intero, anche se su questioni rilevanti per le istituzioni del Paese troviamo punti di incontro e convergenza. Quando li troviamo, dobbiamo salutare positivamente questo risultato e poi continuare nella battaglia politica che ci oppone reciprocamente con lealtà e con la capacità di sapere che ci sono questioni democratiche sulle quali l'unità va ricercata con pazienza e guardando ai beni che sono in gioco e agli obiettivi che si perseguono. In questo caso, l'obiettivo del decreto-legge è l'inizio di una fase di bonifica e di moralizzazione, che deve riguardare gli apparati dello Stato e anche il costume politico di questo Paese.

Fin qui non ci sarebbe nulla di strano, perché ormai è la normalità nei nostri tribunali. Il fatto non normale, o almeno non dovrebbe esserlo nel nostro territorio, è che questo signore, definiamolo così, ha rifiutato il proprio avvocato, dottoressa Alessandra Medde, e successivamente anche l'avvocato d'ufficio assegnato dal tribunale, dottoressa Raffaella Servidio,

concedendo il permesso di riaprire la scuola di via Quaranta, illegale e illegittima sotto tutti i punti di vista, innanzitutto quello della sicurezza (che da solo dovrebbe bastare), ma soprattutto nel merito, perché è una scuola che non segue